Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori per ricordare Roberto Calasso, editore, scrittore e grande intellettuale italiano, scomparso pochi giorni fa. Molta parte delle ultime generazioni è cresciuta sui libri che Calasso, con straordinario intuito, sceglieva e pubblicava con magnifiche copertine color pastello. Nelle difficili vicende dell'editoria italiana, sempre alle prese con i nostri limitati indici di lettura, da sessant'anni spicca il marchio della Adelphi. Ed è stata proprio l'ampiezza degli interessi culturali di Roberto Calasso che ha imposto nel catalogo Adelphi la presenza di testi solo apparentemente eterogenei: di letteratura e poesia; di matematica e storia; di fisica e metafisica; di scienza e filosofia delle antiche culture greca, latina, indiana, cinese e persino babilonese; il tutto nella continua ricerca di quei legami e di quei riferimenti che potevano dare unità e coerenza a una produzione tanto inusuale. Nell'editoria italiana degli ultimi decenni Calasso è stato un *unicum*. È naturale che le case editrici rispecchino la personalità degli editori che le hanno fondate. È stato così con Arnoldo Mondadori, Giuseppe Laterza, Giulio Einaudi, Angelo Rizzoli, Giangiacomo Feltrinelli, Livio Garzanti e Valentino Bompiani: i nomi che hanno dominato la scena editoriale italiana per anni e anni. A questi giganti dobbiamo aggiungere Roberto Calasso, che però, per la qualità e il profilo culturale dell'Adelphi, è stato un caso a sé, e non solo nel mondo editoriale italiano, ma anche nel ben più agguerrito panorama internazionale. Adelphi nasce in quello speciale clima creativo e ideativo dei primi anni Sessanta dell'Italia del secolo scorso. In particolare, nasce dall'incontro, oggi impensabile, di alcune delle più eminenti personalità che hanno fatto grandi gli anni del secondo dopoguerra italiano: la cultura e la profondità di visione di Roberto Bazlen e Luciano Foà, ma anche l'impronta sapiente di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, assieme alla spinta finanziaria di Roberto Olivetti. Da quelle colonne di base è nato quell'intreccio che ha permesso a Roberto Calasso, ancora poco più che ventenne, di far nascere e crescere una casa editrice dove la forza culturale si è sviluppata di pari passo con le regole del mercato. Come è stato detto, Adelphi ha prodotto nei decenni tanti libri belli e i lettori quei libri hanno comprato. Nel mondo editoriale Calasso era in un certo modo un eretico e certamente un solitario. Poteva creare un *best seller* pubblicando l'opera di un autore sconosciuto, ma non ha mai cercato lo *scoop* per vendere, né mai mai ha fatto della classifica dei libri più venduti il criterio delle sue scelte. Si è sempre fidato poco delle correnti culturali alla moda, così come si è sempre tenuto alla larga dalle false culture. Ha costruito Adelphi partendo dall'ispirazione originale di Bazlen e Foà e dalla lungimiranza di Roberto Olivetti. Aveva una capacità ineguagliabile di trovare o inventare autori e temi che lui considerava necessari e che, inseriti nel suo catalogo, lo facevano diventare una grande opera unitaria, dove tutto, anche il diverso e l'opposto, si teneva insieme in un intreccio molto solido di legami e di rimandi. Roberto Calasso è l'autore di quella grande opera culturale collettiva che è il catalogo Adelphi. L'Italia dei prossimi decenni avrà bisogno del successo del Piano di rinascita e resilienza, della vittoria sul Covid-19, di tanti nuovi posti di lavoro e del rafforzamento del sistema economico. Ma la scomparsa di Roberto Calasso ci ricorda che soltanto robuste radici culturali come quelle che lui ci ha regalato

come Ulisse, Roberto Calasso, che ci ha lasciato la scorsa settimana e che oggi giustamente ricordiamo in quest'Aula, è stato molte cose insieme: un uomo dal multiforme ingegno. È stato un formidabile studioso, uno straordinario scrittore, un intellettuale aperto e sensibile, un imprenditore lungimirante, un editore coraggioso, uno scopritore vero di talenti, un innovatore tenace, pur essendo sempre rimasto fedele alla casa editrice, la Adelphi, fondata agli inizi degli anni '60 con Luciano Foà e Bobi Bazlen. A quest'ultimo ha anche dedicato un affettuoso ricordo, con un libro uscito proprio nel giorno della sua scomparsa, dal titolo «Bobi», la cui lettura mi permetto di raccomandare. Come è stato giustamente scritto, Calasso è stato l'ultimo epigono di quell'editoria fatta di e da editori, che in primo luogo ha in mente il libro e che ha come obiettivo ultimo non solo il risultato economico, che pure era conseguito, un vero e proprio programma culturale, nel senso più alto e nobile della parola, quello che si attua proprio attraverso il libro. Così, nel mare spesso tempestoso dell'editoria italiana, Roberto Calasso è divenuto un nuovo riferimento omerico, visto che ha saputo guidare la sua barca, la Adelphi, in modo sicuro, professionale e intelligente verso un porto certo. Calasso ha dato lustro al nostro Paese, che siamo certi non lo dimenticherà.

Signor Presidente, il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione di bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto sono allegate, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa per le entrate e una nota integrativa che espone le risultanze della gestione. L'analisi dei contenuti del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi, sia rispetto all'esercizio 2019, sia rispetto alle previsioni iniziali. Sappiamo bene che a tutte le spese che abbiamo dovuto sostenere per la gestione della pandemia. In particolare, il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019; anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 miliardi. Tale peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali, pari a circa il 6 per cento, e di un significativo aumento delle spese finali di quasi il 40 per cento - colleghi, questo è un dato veramente significativo - è stato determinato dai provvedimenti straordinari e urgenti adottati nel corso dell'esercizio per far fronte alle conseguenze dell'emergenza alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso infatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi approvati dal Parlamento e il peggioramento del saldo, se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore di -78,6 miliardi di euro, è pari a circa 192,3 miliardi 192,3 miliardi di euro. Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale),

Tale situazione si è determinata a causa di un aumento delle spese correnti, pari a +117,4 miliardi di euro, contestuale ad un decremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie, pari a -38 miliardi di euro. Il peggioramento è di oltre 65 miliardi di euro se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario, ovvero la differenza tra le entrati finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso dei prestiti, si attesta nel 2020 a -506,9

- erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in -79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -314.340 milioni di euro per il ricorso al mercato - sono stati progressivamente aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza addottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel complesso, gli scostamenti di bilancio hanno rideterminato i limiti massimi

Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2020, i quali denotano infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive, comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo netto da finanziare - di cui si è detto sopra - discende da una gestione di competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli impegni delle spese finali, pari a 236,8 miliardi di euro in più, e una diminuzione degli accertamenti di entrate finali, pari a -36,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Guardando invece alle entrate complessive - è doveroso farlo - l'entità degli accertamenti, pari a circa 943 miliardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019, per un aumento di 77,5 miliardi di euro, a causa dell'aumento degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti. Dal lato della spesa, la grande crescita degli impegni 2020, sia finali che complessivi, questi ultimi passati da 823,2 miliardi di euro del 2019 a 1.076,1 miliardi di euro nel 2020, è frutto dell'adozione di misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto tra 2020 e 2019, relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si rileva innanzitutto la significativa riduzione degli accertamenti delle entrate tributarie, pari a -33,2 miliardi Nel comparto tributario si registra una considerevole contrazione, rispetto al 2019, delle entrate relative alle tasse e imposte sugli affari, pari a circa - 20 miliardi di euro, che corrisponde quindi

impegni di spesa finali, costituiti dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840 miliardi di euro, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi di euro, raggiungendo un'incidenza sul PIL del 50,9 Tale incremento degli impegni riguarda sia le spese correnti, sia quelle in conto capitale. In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 670,9 miliardi, in forte aumento (117 miliardi) rispetto al così come gli impegni di spesa in conto capitale, che hanno registrato una crescita rispetto al 2019 di 119 miliardi e si sono attestati a 169,2 miliardi. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, in aumento nel 2019 per 16,1 miliardi, gli impegni complessivi di spesa si attestano a 1.076,1 miliardi, con un aumento rispetto a quelli dell'anno precedente per circa il 30,7 Il peso della spesa complessiva rispetto al PIL è passato dal 46 per cento del 2019 al 65,2 per cento del 2020. Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, si rileva che, nell'ambito delle uscite correnti, la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, pari a circa il 55 per cento della spesa corrente. Si tratta in prevalenza di trasferimenti alle amministrazioni locali.

Con riferimento specifico alla dinamica delle spese correnti, si rileva che le categorie che registrano i maggiori incrementi sono quelle relative ai trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni, ai trasferimenti correnti alle imprese, ai trasferimenti in calo gli oneri per interessi passivi, che scendono dai 68,4 miliardi del 2019 ai 66,6 del 2020 - -2,5 per cento, e questo è un altro dato significativo - continuando il *trend* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni, da 49,8 miliardi a 169,2 miliardi - anche questo è molto significativo - riferibile riferibile per 92,6 miliardi alle "Acquisizioni di attività finanziarie" e per 16,4 miliardi ai contributi per investimento ad imprese. Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere, e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui, occorre distinguere quelli provenienti da esercizi precedenti e quelli formatisi nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione).

onorevoli colleghi, questo disegno di legge di assestamento è disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica e ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento, pertanto, riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, le spese - limitatamente alla componente discrezionale gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. A partire dal 2017, il disegno di legge di assestamento è corredato anche da una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza

nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri approvati con la legge di bilancio per il 2021, le variazioni risultanti dalle tabelle annesse all'articolato; l'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 3 della suddetta legge di bilancio, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, disponendo la riduzione per 200 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. In allegato al disegno di legge è anche evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione in termini di competenza e di cassa delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo. Venendo ora all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento in esame insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio con atti amministrativi, unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, come il cosiddetto decreto riordino Ministeri, definiscono le previsioni definiscono le previsioni assestate per il 2021 per le quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta su un valore di -232,8 232,8 miliardi, rispetto a una previsione iniziale di meno 193,5 miliardi, Il peggioramento di circa 40 miliardi è dovuto alle variazioni per atto amministrativo compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di assestamento. In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discende essenzialmente dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni. Essi determinano nel complesso un incremento delle spese finali per oltre 41,5 miliardi di euro. Anche altri saldi evidenziano un andamento negativo. Il risparmio pubblico, e cioè quello dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi, registra un peggioramento di 36,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, anche queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare per 40,6 miliardi, in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali del bilancio, nella misura di 41,5 miliardi di euro, di cui 39 miliardi di incremento delle spese correnti e 2,4 miliardi di incremento di quelle in conto capitale. In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una variazione del saldo netto da finanziare di 1,3 miliardi rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio. Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 1,5 miliardi rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2021. Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento delle stime del DEF 2021 con una contrazione di 461 milioni, a cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di 356 milioni a seguito del monitoraggio degli andamenti effettivi di gettito. Complessivamente si determina una riduzione di 818 milioni. Le entrate extratributarie registrano nel complesso un incremento di 2,5 miliardi, determinato dalla migliore evoluzione, in particolare rispetto alle stime del DEF, delle entrate di alcuni giochi, soprattutto lotterie, e dei dividenti che saranno versati dalle società partecipate. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di credito registrano una contrazione di 120 milioni di euro, interamente imputabile a un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate sempre nel DEF. Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano un aumento di 229 milioni in termini di competenza. Questo aumento è determinato da una maggiore spesa in conto capitale per 315 milioni di euro, a fronte di una diminuzione della spesa corrente (meno 86 milioni di euro) determinata principalmente dalla riduzione di 3.279 milioni della spesa per interessi e redditi da capitale, ma compensata da altre maggiori spese correnti per 3.193 milioni. C'è poi una serie di missioni del bilancio dello Stato che determina una riduzione degli stanziamenti della missione «Debito pubblico», pari a meno 12,5 miliardi di euro, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali a breve termine, di cui non si era potuto tenere conto in sede di bilancio di previsione. In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2021 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 9 milioni di euro derivanti da un aumento delle entrate per 1,525 milioni di euro e da un aumento delle spese finali per 1,516 milioni di euro. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -328 miliardi di euro, con un peggioramento di 52,6 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, ma esclusivamente dovuto alla variazione per atto amministrativo intervenuto nel periodo gennaio-maggio 2021, che ha inciso negativamente sul saldo per oltre 52 miliardi

La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è, per l'appunto, il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate, delle regole e dei criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

presento l'emendamento 1.Tab.2.1, con il quale si propone una variazione compensativa tra diversi programmi di spesa. In particolare, viene incrementata per il 2021 di 744.000 euro la dotazione del programma «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali», e di 56 milioni e di 56 milioni la dotazione del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La copertura di questi incrementi è stata assicurata attraverso la corrispondente riduzione, per 800.000, del programma «Fondi da assegnare», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'emendamento 1.Tab.2.2 propone una variazione compensativa che, per il 2021, incrementa di 40.000 euro la dotazione del programma «Edilizia statale di interventi speciali per pubbliche calamità», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con corrispondente riduzione contestuale del programma «Fondi da assegnare», iscritti nello stato di previsione. Questo incremento andrà a posizionarsi sulla struttura commissariale del sistema idrico Gran Sasso dell'Abruzzo, la cui struttura commissariale abbisognava di questa cifra.

grazie a tutte

Il rendiconto comprende il conto del patrimonio, che evidenzia un peggioramento di 299 miliardi, con un totale di passivo del sistema Italia di 2.215 miliardi.

Le entrate finali sono pari a 569 miliardi e le spese finali a 840 miliardi. Le entrate complessive, che assommano il sistema del debito pubblico, cioè l'estinzione a scadenza e la riaccensione

Il saldo da finanziarie è di 270 miliardi ed è stato finanziato con il debito pubblico. Il risparmio pubblico, che sarebbe la differenza tra le spese correnti meno le entrate tributarie ed extratributarie, è di 105 miliardi in negativo. Dovrebbe essere invece positivo per poter finanziare gli investimenti. Gli interessi passivi sono calati del 2 per cento, ma ammontano a 66 miliardi sul debito pubblico (che oggi è di 2.700 miliardi), perché scontano interessi

o elargizione da parte dell'Europa sono tutto debito pubblico (tutto, perché mi si dimostri che i sussidi sono un'altra cosa). Ci sono, poi, secondo calcoli verosimili,

e ci sono - e la spesa improduttiva. Su questo bisogna puntare: avere certezza e provare a fare delle proposte per venir fuori da questa situazione.

Per l'ambiente ci sono troppe autorizzazioni da richiedere. Il decreto-legge semplificazioni ha fatto dei tentativi, che spero si possano tradurre in pratica, ma l'ostacolo è nella giustizia civile, penale e amministrativa. Pensate che le rocce e le terre da scavo sono ancora considerate rifiuti e se un cittadino, di qualsiasi professione, si permette di trasportare un camion, un trattore o un rimorchio carichi di questo materiale è sanzionabile penalmente, se non ha fatto una pratica che supera di 100 volte il valore della merce. Il Monte dei Paschi di Siena richiederà un'iniezione di denaro pubblico, dopo i 5,4 miliardi già erogati in passato; questo è altro debito che va ad aggiungersi, che secondo me dovrebbe essere addebitato a quelli che l'hanno fatto. Le Autostrade le abbiamo di nuovo incamerate; le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e gli investimenti sono un miraggio. È altresì un miraggio il risanamento dell'Ilva. Con il prezzo dell'acciaio odierno guadagnerebbe molti miliardi, che diventerebbero denaro pubblico, con imposte e stipendi;

che farebbero parte del famoso magazzino fiscale (sono quelli degli ultimi anni). I residui passivi sono 196 miliardi, di cui 105 in conto capitale. Se questi partissero senza vincoli

Noi diciamo invece che l'inflazione al 2-3 per cento aiuta a pagare il debito e questo è un mito da sfatare in Europa. L'inflazione rimescola i fattori della produzione, lasciando indietro qualcuno in qualche fase, ma poi li riprende e dà effervescenza e forza all'economia. Il rendiconto non è perciò modificabile ed è la fotografia dell'Italia al 31 occorra una seria riflessione del Parlamento, della maggioranza così vasta e anche dell'opposizione costruttiva, e sia necessario parlare dei numeri, perché non vedo in prospettiva la volontà di innescare un meccanismo

parliamo di numeri e di azioni che si sono svolte nell'anno 2020, l'anno più difficile che abbiamo affrontato dal Dopoguerra. Un anno che ci ha visti impegnati a prendere decisioni importanti, un anno che ha visto i nostri cittadini dover fare i conti con delle restrizioni, dover vedere le loro attività

da portare avanti per il bene nostro, del nostro Governo e dei nostri cittadini. Ho estrapolato dalla relazione sul

i saldi del rendiconto 2020 registrano un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo del 2019

dai provvedimenti urgenti resisi necessari per affrontare l'emergenza 2020, un anno veramente difficile. Voglio ricordare che la Lega nell'anno 2020 era all'opposizione, ma ha sempre cercato di

però, la nostra voce rimaneva inascoltata e veniva portata avanti, forse, di più la teoria dello «io speriamo che me la cavo», cosa che gli italiani non potevano e non possono permettersi.

che il Covid-19 avesse una soluzione attraverso l'abbassamento dei contagi. Abbiamo avuto una buona estate e la gente ha potuto lavorare, ma poi si doveva affrontare l'autunno. La Lega, a tal riguardo, aveva fatto forti pressioni affinché vi fosse una programmazione dell'autunno, che non è avvenuta. Al contrario, ci si è concentrati sui banchi a rotelle. Abbiamo investito tempo a discutere sull'utilità di questi banchi, che hanno dimostrato di essere, non solo uno spreco di denaro pubblico, ma anche un modo per distrarre.

grazie a tutte

volute credendo fossero efficaci e che, invece, hanno dimostrato la loro totale inefficacia. Mi riferisco anche al reddito di cittadinanza, che è stato, sia pure in un periodo pandemico, di sollievo per i cittadini che non potevano avere il lavoro, ma che, in questo momento, dimostra tutta la sua inefficienza al fine di creare lavoro. L'Italia non può vivere di sussidi. L'Italia deve vivere di lavoro le aziende, insieme ai lavoratori, devono poter produrre per garantire uno Stato certo, che garantisca servizi ai cittadini e che possa, con questi servizi, riuscire a dare risposte anche alle persone più deboli, quelle che hanno sofferto di più in questo anno pandemico. *(Applausi)*.

i dati del rendiconto illustrati dal relatore Pesco sono evidentemente impietosi. Lo stesso relatore afferma che c'è un peggioramento di tutti i saldi. Per qualcuno questo dato è inevitabile e lo è anche per noi. Di fronte all'anno terribile, il 2020, che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia, certamente

Proprio perché questi numeri sono impietosi, dobbiamo riflettere su come è stata gestita l'emergenza, perché gli effetti negativi, per certi versi devastanti, si sono riversati in più direzioni.

il fatto che molte attività sono state costrette a chiudere, non per incapacità imprenditoriali o di coloro che le gestivano, ma perché lo Stato ha chiesto sacrifici e ha imposto chiusure che hanno determinato problemi economici per molte famiglie, non solo per coloro che gestiscono attività, ma per i lavoratori e i dipendenti stagionali e non, che nell'anno 2020, e anche in parte nel 2021, hanno avuto redditi ben inferiori a quelli degli anni precedenti, hanno sofferto e stanno soffrendo ancora a causa della pandemia. Qui oggi registriamo il terzo elemento negativo che riguarda tutti noi: i numeri dei conti pubblici. È ovvio che i malati e le morti hanno inciso nell'immediato sulla vita di tutti noi ed è ovvio che anche le chiusure hanno determinato nell'immediato degli effetti negativi; nel nostro futuro noi vivremo anche degli aspetti preoccupanti legati all'indebitamento che siamo stati costretti a contrarre nel corso del 2020 e del 2021. Sono debiti che si aggiungono a quelli già

che prenderne atto, per un verso; ma dall'altro dobbiamo anche interrogarci se effettivamente gli indebitamenti autorizzati l'anno scorso dall'Europa siano stati indirizzati nella direzione giusta se hanno prodotto i risultati che tutti auspicavamo. Noi siamo convinti che, da questo punto di vista, ci sono grandi critiche e grandi rimostranze Innanzitutto dobbiamo prendere atto del fatto che, ogni qual volta il Governo e il Parlamento adottano provvedimenti di chiusura, gli effetti negativi ci sono e vanno

che non necessariamente hanno effetti positivi sulla salute pubblica, ma che hanno un effetto negativo chiaro sulla vita di tante persone che vogliono lavorare, produrre e mantenere le proprie famiglie.

alcune volte le misure adottate dal Governo precedente non hanno centrato i veri obiettivi e non sono andate nella direzione di dare risposta a tutti coloro che hanno subito dei danni, ma hanno preso direzioni molto discutibili. Lo abbiamo richiamato più volte e diventa forse una litania quella delle opposizioni di allora nel richiamare l'attenzione sui soldi sprecati per i banchi di scuola, con o senza rotelle; però è inaccettabile che, di fronte a un dramma vissuto da tutto il Paese, il Governo precedente si sia permesso il lusso di spendere svariate centinaia di milioni per banchi che ora sono ammassati nei magazzini. Non era certamente quello l'obiettivo

in termini di chiusure e di decisioni che mettono in difficoltà la nostra economia, ma deve essere anche un elemento di allarme per il prossimo bilancio. È ovvio che la prossima legge di bilancio sarà forse uno degli degli appuntamenti più difficili per questo Governo, perché le politiche economiche di partiti così diversi non possono che trovare difficoltà nel far emergere un testo e una legge di bilancio comune tra PD, MoVimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e LEU, che hanno visioni economiche molto distanti e profondamente diverse. Questa sarà la vera sfida dei prossimi è evidente che non potremo condividere la mentalità più negativa di questi partiti, che riguarda ad esempio la tassazione. le tasse siano una cosa bellissima, non riteniamo che la priorità del Governo sia applicare una tassa di successione e quindi non condividiamo le impostazioni del segretario del PD, Enrico Letta, così come non condividiamo la mentalità la mentalità del MoVimento 5 Stelle, secondo la quale solo attraverso il reddito di cittadinanza universale si possano sollevare le sorti del Paese. Crediamo nella cultura del lavoro e crediamo che che aumentare le tasse non significhi avere più entrate, ma il più delle volte significa averne meno, perché si fanno fallire attività e aziende. Chiediamo quindi che, nel prossimo futuro, questo tipo di approccio venga preso in considerazione e sia il perno dell'azione del Governo nella redazione della legge di bilancio, perché solo attraverso la riduzione delle tasse

la Lega, in questo caso, sosterrà la sua azione fino alla fine

Il rendiconto è sostanzialmente inemendabile ed espone le risultanze contabili così come sono, però ci offre una fotografia puntuale e precisa della situazione. La legge di assestamento, invece, ci aggiorna sugli stanziamenti di bilancio e accerta la rendicontazione dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Dall'attenzione che c'è su questi argomenti, vediamo che è materia arida, che non entusiasma nessuno. Cercherò allora, se ci riesco, di traslarla nel mondo dell'economia reale. È come se oggi ci trovassimo nell'assemblea dei soci, chiamati ad approvare il bilancio dell'anno precedente. Per una società di capitali non è un'assemblea banale, è l'assemblea più importante, perché è quella che

un ombrello dal punto di vista economico, nel senso che ci ha permesso di sforare tutte le previsioni che avevamo fatto. Siamo andati oltre lo sforamento del debito,

che un'azione demagogica che non risolve il problema, o quota 100 - che non hanno centrato gli obiettivi. Colleghi, prima o poi dovremo avere la forza ed il coraggio di analizzare fino in fondo Ci sono realtà economiche territoriali, come il settore del turismo, che non trova personale stagionale perché la gente sta a casa per poter prendere il reddito di cittadinanza.

la filiera turistica sta soffrendo tremendamente di questo fenomeno, rendiamocene conto. Si tratta di stabilire che chi gode del reddito di cittadinanza e stipula un contratto di lavoro stagionale

Il presidente Draghi ha parlato di debito buono e di debito cattivo. Nel 2020 abbiamo fatto solo debito cattivo, i dati lo testimoniano e lo confermano. Il debito buono è quello che va negli investimenti e gli investimenti sono fermi. Abbiamo però - ecco l'ombrello - i fondi del PNRR,

troppo tardi. I progetti di cui al PNRR devono essere messi a terra entro il 2026, ma siamo ancora lontani dall'individuazione puntuale di quanto dobbiamo fare. Spero molto nell'attività

ma è anche la relazione del collegio sindacale, che è l'organo di controllo. E chi è l'organo di controllo del bilancio dello Stato? La Corte dei conti, che rilascia il cosiddetto giudizio di parificazione, che in pratica è la relazione del collegio sindacale che conferma ai soci il buon andamento dei numeri che sono scritti. Non

banalizzando, non sappiamo se i numeri che abbiamo indicato sono proprio quelli veri, perché non si riesce ad avere contezza esatta

poco fa e sicuramente lo riprenderà il mio Capogruppo in Commissione bilancio, senatore Damiani, nella sua dichiarazione di voto. Noi vogliamo che il Governo

Poniamo mano in maniera seria e precisa a quelle riforme che non hanno centrato l'obiettivo: mi riferisco a reddito di cittadinanza e quota 100 che non hanno raggiunto l'obiettivo per il quale erano state

il suo appoggio perché ci sia veramente un cambio di passo veloce e rapido per far ripartire il Paese. Nel frattempo è arrivata la sesta medaglia d'oro e credo che questo sia un ottimo auspicio perché il futuro sia migliore.

del Governo, oggi siamo qui a discutere di un argomento che poco appassiona

Quest'anno il rendiconto e l'assestamento risentono di quella crisi sanitaria, economica e sociale da Covid-19 che ha colpito il mondo intero e in modo particolare l'Italia. Il rendiconto è una fotografia della gestione dell'anno che si è concluso, il risultato di quel disastroso 2020 in cui, a fronte di un PIL che si è vistosamente contratto anche a causa delle chiusure,

viziati dai codici Ateco, per carità, per aiutare la cittadinanza anche attraverso gli enti locali. Infatti, si rileva che nell'ambito delle uscite correnti la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, pari a circa il 50,5 per cento della spesa corrente. Si tratta, quindi, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali e a enti previdenziali (la cassa integrazione).

eravamo all'opposizione. Vorrei infatti ricordare che la Lega non si è mai sottratta dall'approvare gli scostamenti di bilancio che si sono susseguiti, salvo poi essere molto critica sullo stanziamento delle risorse deliberate. Vorrei ricordarvi, colleghi, che nel 2020 abbiamo deliberato più di 200 miliardi di scostamento, abbiamo inserito spese

i soldi che stiamo aspettando dall'Europa e che dovrebbero caratterizzare gli investimenti per i prossimi cinque anni, non arrivano a 200 miliardi, sono 191,5.

è stata gestita in modo inadeguato. Ricordo che il 2020 è stato l'anno dei DPCM di Conte, della gestione imbarazzante del commissario Arcuri,

forse migliore, ma in cui solo noi della Lega chiedevamo se saremmo stati pronti per l'ondata dell'autunno. Vengo così all'argomento che più mi sta a cuore, ossia evidenziare se si poteva fare di meglio. A mio avviso sì. Non sono un medico, ma sono abituata ad approfondire e guardare i dati e già nel maggio 2020 seguivo con attenzione il lavoro di quei medici che, in scienza e coscienza, avevano semplicemente pensato di curare il Covid. Nel maggio 2020 i medici di Ippocrate, i medici delle cure domiciliari e l'assessore Icardi della mia Regione, il Piemonte, avevano già individuato quella che dovrebbe essere la cosa più naturale per un medico,

Quella vigile attesa che, secondo me, ha portato a tanti, troppi ricoveri (e ne ho degli esempi), talvolta con esito purtroppo fatale. Si poteva fare molto meglio. Nell'autunno 2020 si poteva iniziare a curare le persone, mentre si è scommesso su un'unica strategia. C'è stata una vigile attesa dell'arrivo del vaccino, quando avremmo potuto invece contrastare l'ondata autunnale semplicemente curando. tutto ciò c'entra con il rendiconto. Eccome se c'entra. Il disastro economico dovuto alle chiusure è da attribuirsi in parte anche a una visione miope sul fronte delle cure. Questa è la mia opinione. Il nuovo Governo, con la sua ampia maggioranza, ha ereditato la situazione sanitaria esistente, una campagna vaccinale disorganizzata e partita male, che sicuramente è riuscita a ricevere impulso grazie all'operatività e alla capacità del generale Figliuolo, uomo abituato a raggiungere gli obiettivi. Il ministro Speranza è rimasto e anche ultimamente però, ha dichiarato che la vaccinazione è l'unica arma a disposizione per combattere la pandemia.

tutti i colleghi *(Applausi)* anche sui piccoli problemi. Forse sembrano piccoli - parliamo di 40.000 euro - ma in realtà la struttura ha bisogno di questa possibilità per poter operare al meglio.

un passo in avanti. Mi auguro che nei prossimi provvedimenti questi pochi fondi - ripeto, si tratta di 40.000 euro - possano essere davvero destinati all'utilizzo per il quale sono stati indicati oggi nel provvedimento in

Signor Presidente, non posso che ringraziare tutti i colleghi e le colleghe intervenuti, a partire dal collega Ferro alla collega Di Girolamo, Ferrero e tutti gli altri, perché hanno dato sicuramente degli spunti interessanti per riuscire a migliorare la nostra attività, sia come Commissione bilancio, sia anche per la supervisione e il controllo dei conti pubblici. È stato ricordato l'apporto dato dalla Corte dei conti, che ogni anno ci fa capire dove può essere migliorato il controllo e le cose che vanno sistemate. Ogni anno, infatti, c'è qualcosa che non va nei conti pubblici, la Corte dei conti ce lo fa presente e il Governo dovrebbe impegnarsi

e soprattutto anche - aggiungo io - per la tutela del paesaggio e della rete infrastrutturale verde. Sarebbe veramente molto utile e lo faremo sicuramente attraverso i fondi che verranno erogati attraverso il PNRR già da quest'anno. L'impegno della Commissione bilancio - ma penso di tutti i colleghi - è quello di fare in modo che questi soldi vengano impegnati e spesi nel più breve tempo possibile, logicamente mantenendo quei presidi utili affinché non vengono sperperati e utilizzati in modo non idoneo.

l'evoluzione della situazione economico-finanziaria del Paese, nel proprio intervento hanno chiaramente esplicitato anche la preoccupazione. Nessuno di noi si aspettava una malattia di questo tipo; nessuno di noi si aspettava la necessità di dover intervenire con provvedimenti così importanti per cercare di tamponare situazioni deficitarie, preoccupanti e che erano allo stremo. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che una malattia del genere avrebbe potuto scoperchiare anche i vasi tenuti chiusi da molti anni,

dovremo farne tesoro tutti, dovremo imparare dagli errori del passato e da quello che stiamo vivendo quotidianamente e che dovremo vivere ancora. Dovremo farne tesoro anche nella stesura della legge di bilancio, perché sarete tutti chiamati a dare il vostro contributo, anche se adesso vi sembra una prospettiva lontana e sembrano più vicine le vacanze e le spiagge. Ci sarà un momento in cui si rientrerà e improvvisamente caleremo tutti la testa verso questi conti, perché poi dovremo

Prendo atto anche delle considerazioni che sono state fatte sul rendiconto, che peraltro è un provvedimento chiuso, senza possibilità di modifiche. Voglio ricordare che le proposte di assestamento determinano in generale un miglioramento del saldo netto da finanziare per 1.300 milioni in termini di competenza e sono sostanzialmente neutrali in termini di cassa. Le variazioni complessive determinate da queste proposte di assestamento sono sostanzialmente neutrali anche in termini di indebitamento delle pubbliche amministrazioni. Va anche tenuto presente che questo provvedimento recepisce, per 41,55 miliardi in termini di competenza e per 52,48 in termini di cassa, gli effetti delle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi adottati in corso di anno. Voglio ricordare, in particolare,

per il quale, peraltro, il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento. Voglio anche segnalare che questo è il secondo anno che per l'assestamento presentiamo una relazione tecnica

dicevo, ci tengo a segnalare che per il secondo anno, l'assestamento presenta una relazione tecnica che dà maggiore trasparenza dei dati, con riferimento all'assestato del conto e con un raccordo col saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, le previsioni assestate, il conto della pubblica amministrazione tendenziale e anche il 2021 assestato. alle entrate, sottolineo che i 2,3 miliardi che sono stati inseriti in attestamento sono molto importanti, perché sono stati destinati a interventi di contrasto degli effetti negativi generali della pandemia.

da tutti i Gruppi parlamentari - e, in materia di istruzione e emergenze nazionali, indennizzi per i risparmiatori, per l'edilizia scolastica e la ricostruzione delle aree terremotate. Voglio ringraziare, infine, la Commissione bilancio, che mi vede impegnata praticamente tutte le settimane. Voglio ringraziarla per la collaborazione e per l'attento esame che sempre fa su tutti i provvedimenti, anche su questi, che sono un po' aridi e che però, in effetti, danno conto della situazione vera del Paese.

Signor Presidente, il complessivo peggioramento dei conti pubblici, con una diminuzione delle entrate finali pari al 6 e un significativo aumento delle spese finali di quasi il 40 per cento, è naturalmente il prodotto delle misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza pandemica. Queste misure e i vari scostamenti di bilancio per finanziarle hanno portato il saldo negativo dai 78 miliardi di euro delle previsioni iniziali a più di 192 miliardi. Si può continuare citando i dati del comparto tributario, con numerosi settori che hanno segnalato una contrazione a doppia cifra e parlando del maggior ricorso al mercato finanziario o della diminuzione delle entrate extra tributarie e così via. un quadro letteralmente terremotato rispetto alla fase pre-pandemica; un quadro anche difficile da definire per la sua rapida evoluzione, come in qualche modo ha notato anche la Corte dei conti, quando ha ricordato che diverse entrate tributarie poste in previsione in realtà sono collegate a variabili di natura macroeconomica, motivo per cui non sempre sono calcolabili con esattezza. In fondo, questa difficoltà è una costante dei conti pubblici. Tuttavia, nel contesto nel quale ci muoviamo, questa criticità può rivelarsi esplosiva, se le previsioni di crescita non verranno mantenute. È un dibattito che in Commissione facciamo dal primo scostamento di bilancio. Ci apparve subito chiaro che ci incamminavamo su un sentiero che avrebbe gonfiato a dismisura il nostro debito pubblico e, per non farlo cadere addosso alle prossime generazioni, non serviva e non serve solo un grande impegno: serve soprattutto un cambio di mentalità rispetto al modo con cui, in troppe fasi della storia, l'Italia ha gestito le sue finanze. non c'era un'altra strada all'indebitamento, senza il quale - l'abbiamo intravisto nella crisi dello scorso decennio - l'economia sarebbe entrata in una spirale depressiva senza possibilità di ritorno. Ma oggi non c'è altra strada che quella di una crescita sostenuta, con un'Italia che, alla fine della pandemia, si attesti finalmente sopra la media europea, superando, cioè, quei limiti e quei ritardi strutturali che ne hanno determinato, negli ultimi una crescita più debole, anche durante cicli economici favorevoli. Oltre alle risorse del *recovery fund*, tra cui la cospicua parte a fondo perduto, non dimentichiamoci che abbiamo due elementi a nostro favore, ma che tali potrebbero non essere per sempre: il cappello della Banca centrale europea e la sospensione del Patto di stabilità. Certo, sarebbe folle se l'Europa tornasse alla stagione e alle regole di prima; ma sarebbe altrettanto folle pensare che la BCE possa fare per sempre incetta di titoli sui mercati per finanziare il nostro debito e tenere bassi i tassi di interesse. Cosa succederà il giorno in cui i tassi torneranno a crescere, se noi nel frattempo non ci saremo dotati di una crescita in grado anche di accompagnare la riduzione del debito? Credo, quindi, che questi numeri e che questi provvedimenti, che a volte vengono affrontati un po' stancamente dal Parlamento, dicano tutto sulla responsabilità che dobbiamo avere nella gestione degli aiuti europei, nelle misure per arginare la quarta ondata, nella messa in campo di riforme che aiutino il Paese a sconfiggere le sue antiche fragilità, da quella della giustizia a quella del fisco, dalla concorrenza al codice degli appalti, che saranno le grandi questioni di settembre. Lo ripeto ancora una volta: non è questo il momento delle divisioni e delle bandiere di parte; è ancora il momento dell'unità nazionale, delle scelte anche impopolari, se queste servono per costruire l'interesse generale delle generazioni presenti e soprattutto di quelle future. È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

hanno subìto a seguito dello *shock* pandemico dal febbraio 2020. La situazione ha riguardato il mondo intero e ha riguardato molto pesantemente anche la nostra Italia. I senatori della Commissione bilancio, che da diciotto mesi lavorano sui numeri, sui provvedimenti, sugli scostamenti e oggi, appunto, sul rendiconto e sull'assestamento, hanno la responsabilità di dire in quest'Aula che la situazione è, sì, sostenibile, ma anche che l'Italia non ha più la

La spesa per interessi non aumenta molto, rimane ferma al 3,5 per cento del PIL, ma questo grazie a una situazione di tassi di interesse pari allo zero o negativi che non possiamo sicuramente attenderci che continui in futuro. Presidente, anche le entrate totali si sono fortemente contratte, naturalmente soprattutto quelle correnti, per via della contrazione e della chiusura di molte attività, che hanno avuto pesanti ripercussioni soprattutto sulle entrate tributarie, le imposte dirette in particolare. Le uscite totali, sia correnti che di capitale, hanno registrato un forte aumento: qui voglio soffermarmi, perché le integrazioni salariali, gli assegni, i sussidi assistenziali, ma anche, sul fronte delle imprese, le garanzie a fronte di finanziamenti alle imprese e i contributi a fondo perduto costituiscono un'operazione di salvataggio dell'economia che però ha uno stampo di assistenza che né i conti pubblici, né la filosofia politica che noi sosteniamo possono permettersi di perpetrare in futuro. Il futuro può essere solo costituito da lavoro e da crescita e questo lo attesta il rendiconto 2020. Molti colleghi hanno confermato saldi e numeri, però va rimarcato che tutti i saldi registrano un peggioramento: il saldo netto da finanziare è a oltre meno 263 miliardi; il risparmio pubblico, sia con riferimento all'anno precedente, sia con riferimento alle previsioni iniziali, registra un netto peggioramento. al ricorso al mercato finanziario, il rendiconto ci dice che il soccorso all'economia e alla società ha lasciato ampie tracce che vanno risanate. risanate. L'assestamento - noi lo sappiamo - assolve il compito di apportare delle variazioni allo stanziamento di bilancio. Le variazioni di bilancio, assieme alle variazioni apportate fino al 31 maggio dagli atti amministrativi dei provvedimenti legislativi, costituiscono le previsioni assestate. Anche in questo senso vediamo un netto peggioramento dei saldi: un peggioramento

di interventi che hanno reso difficili i nostri conti pubblici, come quota 100 o il reddito di cittadinanza, misure che sicuramente non hanno funzionato come si voleva e che devono essere riviste, l'assestamento 2021 ci consegna una speranza per il futuro e delle misure che possono innestare una crescita. È evidente che la situazione attuale necessita di vie d'uscita e la via di uscita è una e si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma perché tale Piano sia efficace, serve che la strategia che il Governo ha posto in essere per risanare i conti pubblici e riportare il debito pubblico verso un obiettivo di medio termine, basandosi sulla crescita,

del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 2026 (e voglio sottolinearlo: entro il 2026), ma, tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, noi dobbiamo attivare quei 1800 miliardi di risparmio privato che devono contribuire allo sviluppo, alla crescita e all'attuazione delle riforme. Poi, naturalmente ci sono le riforme. Una stagione molto difficile, che sana gli ultimi venti anni di mancate riforme. La riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione le abbiamo già approvate. Stiamo faticosamente portando a termine la riforma della giustizia penale e della giustizia civile; poi avremo quella della concorrenza e del fisco.

che ci sia stabilità, non solo in questa legislatura, che deve concludersi con una sorta di unità nazionale, ma che ci sia stabilità fino al 2026 e oltre. Noi dobbiamo riconoscere che abbiamo visto delle stagioni veramente dispendiose, in termini di serietà e in termini di tempo, con dei diversivi populisti e con un gioco delle parti davvero sterile, che sicuramente non aiuta l'Italia. Pertanto, nel dichiarare il voto favorevole di Italia Viva al rendiconto generale e all'assestamento di bilancio, io auguro veramente, a ciascuno di noi e a coloro che arriveranno dopo di noi, di saper portare con grande serietà il peso di questa grande responsabilità e di questa bellissima sfida.

l'economia e la finanza del nostro Paese. Ritengo sia giusto partire da un numero, quello che rappresenta, per quanto riguarda l'esercizio 2020, il saldo netto da finanziare: negativo Se poi guardiamo al saldo netto da finanziare per il 2021, nell'assestamento, il dato peggiora ancora, perché andiamo oltre i 300 miliardi. miliardi. Io non mi stupisco, ovviamente. Dall'opposizione, noi di Fratelli d'Italia non siamo qui per fare populismo e demagogia, né per sparare contro qualcuno. Capiamo che questi numeri vanno letti nell'ottica della crisi pandemica e degli interventi straordinari, che ci sono stati e che dovevano esserci.

ritengo sia doveroso, e sia addirittura un obbligo di coscienza per un parlamentare e per un amministratore, interrogarsi sul fatto che, mentre indebitiamo il nostro Paese e i nostri figli, quel denaro sia speso in modo efficiente ed efficace, che quel denaro non sia sprecato, che quel denaro non costituisca una continuità su proposte, fatte da alcune forze politiche, anche in piena onestà intellettuale, che poi si sono dimostrate errate. Quindi, cari colleghi, e mi rivolgo a tutto l'emiciclo, sarebbe ora di interrogarsi sul fatto che, 2021, 15 miliardi sono impegnati e - mi permetto di dire - sprecati nel reddito di cittadinanza

su questo spreco di denaro pubblico. Un conto infatti sono le misure emergenziali, un conto è operare in modo straordinario su coloro che necessitano di un reddito di di emergenza; altro conto è mantenere in modo strutturale un reddito, quello di cittadinanza, che non ha nulla a che vedere con lo sviluppo del Paese. Oggi due quotidiani nazionali (non uno, ma due), gli unici due quotidiani economici nazionali, di fatto sparano sul reddito di cittadinanza. Lo fa «Italia Oggi», con un imprenditore che ha scommesso sul nostro Paese, sul Sud, e che dice che con il reddito di cittadinanza non si trovano lavoratori. Le stesse cose le dice Confagricoltura, le dicono i coltivatori diretti (Coldiretti) e le lamentano gli imprenditori del mondo alberghiero e turistico. Io provengo da un territorio, da una Provincia e da una Regione che vivono di turismo. E il turismo lamenta che non si trovano più lavoratori da quando c'è il reddito di cittadinanza. Ci sono quindi i coltivatori diretti, gli agricoltori, gli imprenditori del turismo;

E noi perseveriamo nel pagare chi non lavora, chi - lo dice il presidente dell'INPS Tridico, cari colleghi - non ha prospettive di occupazione! Spesso queste persone sono volontariamente e strutturalmente fuori dal mercato del lavoro. Due terzi dei 3.700.000 percettori del reddito di cittadinanza nel 2018 e nel 2019 non erano iscritti nei registri dell'INPS. Tridico, presidente dell'INPS, ha certificato la non occupabilità di queste persone. di una misura che impegna 15 miliardi su due anni, di un assistenzialismo che ha dimostrato di non poter avere in sé quelle politiche attive con le quali nella fase iniziale dell'approvazione, a inizio legislatura, voi giustificavate il reddito di cittadinanza. Ebbene, a tre anni di distanza le politiche attive sono inesistenti, nell'ambito di tutto quello che è il teorema sul reddito di cittadinanza. un assistenzialismo senza lavori socialmente utili, perché un cittadino, cari colleghi, si aspetterebbe che colui che prende soldi senza lavorare vada almeno a pulire le piazze del paese, a ripulire i parchi, ad assistere gli anziani, a fare lavori socialmente utili. Non è accaduto nulla di tutto ciò, al di là delle intenzioni.

Ma magari aiuta invece i delinquenti usciti di galera, i lavoratori delle mafie e delle camorre, che risultano nullatenenti e che con quei soldini ci comprano le sigarette, perché magari sono abituati a introitare migliaia di euro illegali al mese (e si prendono anche il reddito di cittadinanza). Ecco l'etica sbagliata, che non può essere accettata nel momento in cui il nostro bilancio piange per i numeri che or ora ho detto.

in futuro, vorrei vedere maggiori investimenti veri nel nostro Paese; maggiori investimenti ad esempio, proprio perché noi crediamo nel sociale, per l'estensione degli ammortizzatori sociali. È lì che io vorrei vedere nel rendiconto 2021 quello che avremo tra qualche mese; oppure vorrei vederlo anticipatamente nella NADEF. Vorrei vedere davvero lì gli ammortizzatori sociali che diventano un patrimonio della comunità italiana tutta, dall'artigiano al commerciante, dal dipendente al parasubordinato. Vorrei vedere maggiori investimenti, che - ahimè in tema di Covid. Dove sono, nel secondo giro della pandemia, gli interventi e gli investimenti sui trasporti, gli investimenti sui trasporti, sulla scuola e sulla medicina territoriale? Pensate davvero, colleghi, di risolvere tutto solo con il *green pass*? Pensate davvero che obbligare un cittadino o un ragazzino che va a scuola ad avere il *green pass* voglia dire risolvere i problemi del Covid? No! Investite e investiamo, utilizziamo bene il debito, con la sanificazione dell'area delle scuole e con l'intensificazione, in termini quantitativi, dei trasporti!

poco o nulla. Anticipo infatti, colleghi, che la riforma fiscale, che ci avevano promesso per fine luglio, non arriverà neanche a fine luglio del prossimo anno. Non ce l'avremo, perché non è prevista negli investimenti. Con 3 miliardi di euro non si fanno riforme fiscali: è una presa in giro!

tutti i grandi pappagalli dell'*austerity*? Dove sono finiti coloro che ignoravano la legge di Kaldor-Verdoorn sulla produttività, in rapporto alla crescita economica del Paese?

Presidente, diversamente dal collega che mi ha preceduto, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare del quale sono espressione.

proponendo sin da subito una domanda, come fanno gli avvocati penalisti in aula: se non ci fosse il giudizio sul rendiconto, cosa sarebbe la dimensione politica sull'attività gestionale delle risorse e dei documenti contabili? Sarebbe immaginabile un'attività di valutazione politica e di gestione della responsabilità politica, senza esprimere una valutazione sui documenti contabili del nostro ordinamento? Assolutamente no! Saremmo uno "scritturificio" di virtù, senza nessuna verifica a valle. Ora dobbiamo verificare e i colleghi che mi hanno preceduto, a partire dai due relatori, la senatrice Faggi e il senatore Pesco, hanno messo in evidenza quali sono i numeri indiscutibili della gestione contabile. Voglio rendere volgarizzata questa materia, ovvero non volgare, ma comprensibile a tutti. È immaginabile la gestione delle risorse finanziarie ed economiche, senza usare l'istituto dell'assestamento, dell'accertamento dei residui attivi e passivi? Assolutamente no e questo perché non stiamo parlando del conservatorio di musica «Luisa D'Annunzio» di Pescara, della gestione dell'ordinamento statuale, che si fa carico anche di emergenze di portata nazionale, come la pandemia. È questo il tema che deve indurre tutti ad essere ragionatori, ragionevoli (non idioti, si sarebbe detto nell'antica Atene, Atene, intendo non quelli condannati per mancanza di mente, ma coloro i quali sbagliavano le proporzioni nella misurazione, non considerando i fatti del contesto). Il fatto prevalente del contesto è questa rottura di civiltà che si chiama pandemia, che è più di una crisi ciclica, ed è chiaro che questo porta con sé il debito, l'indebitamento qualificato come debito buono, poiché cerca di sostenere la vita e la ruota dell'economia che deve ricominciare.

A pagina 8 della requisitoria orale del procuratore generale della Corte dei conti Canale, si mette in evidenza che la gestione è meritevole di voto favorevole, ma ci sono aspetti che vanno corretti e messi in evidenza. Si dice

come l'ingresso della contabilità di ANAS nel perimetro riservato della gestione non sottoposta al patto di stabilità. Non è un gioco di parole, né un prestito che prendo da registri Buffetti: se l'ANAS potesse contare sulla gestione delle risorse finanziarie al pari delle Ferrovie dello Stato, avrebbe velocità e flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi. Si chiamano risorse normative,

fare in modo che tutti i cespiti del demanio dello Stato vengano rubricati, in quanto devono produrre virtù finanziaria ed economica

34.000 soggetti partecipati creano affanno anche nella redazione dei documenti contabili. È per questo che ci serve un lavoro di merito premuroso, che non venga vinto dall'ideologia o dal dibattito emotivo di parte. Voglio anche evidenziare, ad esempio, che financo il Ministero della giustizia è oggetto di appunto,

non è un adempimento burocratico, ma l'adempimento che consente ai rappresentanti della Nazione di esprimere una valutazione. Nella filosofia morale, la valutazione evoca l'etica. Nella gestione contabile, la rendicontazione è l'etica applicata alla nostra responsabilità. Servono informazioni, dettagli, contabilità analitica. Nel progetto di opera pubblica non è il segno, il colore, a fare l'anima del progetto, ma il computo metrico. Nella gestione delle risorse finanziarie è esattamente il dettaglio analitico che consente il giudizio consapevole, altrimenti diventiamo come elementi di arredo, che va sempre bene, ma non è necessario. È su questo, allora, che invito ad acquisire una consapevolezza che determini anche un giudizio di merito attrezzato, responsabilizzato, che poi fa sì da curvare, quando serve, anche la correzione del cammino delle risorse. Quando nel Novecento migliore si selezionavano coloro i quali si candidavano, Paolo De Ioanna spiegò, in una bellissima giornata destinata alle giovani generazioni, che le risorse sono quelle finanziarie (ce ne stiamo occupando); quelle normative (che produciamo quando ci raccogliamo); poi ci sono quelle tecnologiche tecnologiche e, importanti, quelle di visione strategica, che consentono di cucire quanto si mette in campo sul piano dei beni limitati, che sono le risorse finanziarie, con i beni illimitati, che sono le idee. Servono le idee per fare in modo che la misurazione sia all'altezza della sfida. Siamo stati chiamati a una sfida più grande della nostra previsione, per questo l'intervento del collega va bene, però è collocabile, quasi come un loculo, in una posizione di parte. Serve invece la presa di coscienza della straordinarietà dell'accaduto. Per queste ragioni, queste ragioni, intervengo per sostenere il lavoro che è stato fatto dall'ordinamento e mi viene quasi da dentro l'emotività che, davanti alle rotture di civiltà, dovremmo essere oltre l'unitarietà, a livello di univocità dei punti di vista. Per questa ragione, il Gruppo PD mi ha incaricato di dichiarare il voto favorevole.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito i numeri. Siamo in una fase di peggioramento dei saldi e in una situazione assolutamente straordinaria,

oltre ai dati fondamentali del rendiconto (che è uno strumento decisivo, per quanto misconosciuto anche nella nostra discussione), si facesse una valutazione *ex post*

per rendere più equo, giusto e sostenibile il lavoro di sostegno e aiuto a famiglie e imprese.

politiche capaci di dare una risposta occupazionale. Tuttavia, non è certo il reddito di cittadinanza a

astratto - su ciò che funziona e ciò che non funziona, nonché su cosa devono essere le nuove politiche attive per il lavoro, a partire dalla leva della formazione,

dico "noi" genericamente - abbiamo distrutto la formazione tecnica e questo è il primo problema in relazione al rapporto con le politiche attive del lavoro. Insomma, colleghi e colleghe, penso che, se cominciassimo a fare un discorso di merito che va oltre il posizionamento, forse daremmo un contributo. Il secondo grande tema la sanità. Fatemi dire una cosa: ma voi siete contenti - io no - che l'Europa abbia deciso e fatto un contratto con il quale si aumentano i costi di Pfeizer e Moderna? Io no,

a proposito della riforma del sistema sanitario, ci troveremo in emergenza non solo sui vaccini - e dobbiamo avere la consapevolezza che saremo

(RNA) è una grande rivoluzione nel sistema sanitario della farmacologia, che affronterà i temi della vita. Come gestiremo queste partite? Insomma, c'è una grande sfida che richiede un salto di qualità, dal punto di vista della cultura politica di tutti noi, considerino i problemi non solo oggi, non solo alla ricerca del *tweet* o dell'applauso, ma con una visione e una strategia. Senza di questo, non andremo da nessuna parte.

la situazione imprevista in cui si è trovato in quest'anno il Paese. Abbiamo affrontato un'emergenza sanitaria importante. Il 2020 è stato l'anno della chiusura

quindi una situazione straordinaria, affrontata con strumenti straordinari. È per questo che nel corso dell'anno siamo dovuti intervenire più volte, anche modificando

ci deve responsabilizzare. Proprio perché siamo andati su questa strada obbligata e stiamo indebitando le future generazioni, oggi dobbiamo essere

adesso alle spalle il debito cattivo, e pensare solo eventualmente a quello buono, perché i numeri sono comunque drammatici. Voglio soltanto ricordare come il bilancio dello Stato sia cresciuto dagli 870 miliardi del 2019 ai 1.150 del 2021. Questi dati ci fanno ben capire come oggi le spese fini a se stesse non siano più possibili nel Paese, mentre dobbiamo andare esclusivamente sulla strada degli investimenti e della modernizzazione.

che questi numeri impongono una decisa presa di posizione e l'unica cosa, come dicevo, è quella di fare le riforme: in testa a tutte c'è la battaglia delle battaglie, la riforma fiscale *(Applausi)*, perché non ci può essere oggi crescita del Paese, se non abbassiamo le tasse alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, che sono il volano della nostra economia, e su questo Forza Italia da tempo è impegnata. È l'unica strada oggi per portare il Paese fuori

a dire che i risultati non sono venuti, perché oggi la pandemia ci ha messo di fronte veramente tante situazioni, ma qualcosa la crisi ce l'ha insegnato.

siamo d'accordo sulle misure di contrasto alla povertà, che però sono altro e vanno tracciate più su una linea di politiche attive del lavoro e non, come dicevamo, di assistenza fine a se stessa. Altro tema dolente, che sicuramente si riscontra dai dati di bilancio, è il pagamento in favore delle imprese dei debiti della pubblica amministrazione. Dobbiamo fare di più.

per i diritti dei nostri cittadini, ma perché oggi costa tanto allo Stato. Quindi, anche la riforma della giustizia va nella direzione dello sviluppo

ma sono simbolo e sintesi di scelte che determinano il futuro della nostra comunità e soprattutto la qualità di ciò che vogliamo realizzare per noi e per i nostri figli.

Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento questi risultati, dai quali evinciamo gli effetti di tutta la spaventosa realtà provocata dalla pandemia. Lo voglio ricordare: tutto è partito con la dichiarazione dello stato di emergenza il 31 gennaio dello scorso anno; il primo stanziamento pensato era stata l'anticipazione del 66 per cento sul fondo di solidarietà ai Comuni, che sono stati gli enti in trincea. I sindaci, infatti, sono stati coloro che, rischiando con le proprie decisioni, hanno cercato di dare risposte ai cittadini e agli imprenditori sul territorio, che, terrorizzati, non sapevano dove andare né cosa fare, ma soprattutto

iniziava a fare vittime e a espandersi nel cuore della Lombardia e del Veneto, a Codogno e a Vo' Euganeo, quando abbiamo mandato

dovrà fare assistenza al monitoraggio dell'avanzamento finanziario e procedurale degli investimenti pubblici, per la mappatura del portafoglio di progetti finanziati in ottica programma-progetti, per la ricognizione di aree e progetti in criticità realizzativa da sottoporre ad azioni di supporto: che il Signore ci aiuti, ma andiamo oltre. La Lega ha comunque sempre avuto, anche dai banchi

Ricordo che la Lega non si è tirata indietro rispetto all'approvazione degli scostamenti, perché era necessario, bisognava farlo.

invece la Lega continua a starci, perché ritiene che in questo momento si debba fare un passo indietro rispetto ai propri ideali di partito;

per rispetto ai nostri cittadini, alle nostre imprese, ai nostri commercianti e alle nostre famiglie.

Ora abbiamo la possibilità di vedere cosa non ha funzionato e cosa si può fare per migliorarlo e renderlo più efficiente. Bisogna fare in modo che gli aiuti arrivino, sì, alle persone che non hanno altro modo di sostenersi, ma non è pensabile che venga dato il reddito di cittadinanza a persone che già *ex ante* non hanno diritto ad averlo.

Soprattutto non chiudiamo gli occhi davanti al fatto che i progetti di utilità collettiva (PUC) non hanno funzionato, come ci hanno riferito i rappresentanti di ANCI. Non hanno funzionato, perché la formazione che si è cercato di fare non ha avuto successo, in quanto il livello è mediamente molto basso e quindi non si riesce ad impiegare queste persone.

modo. Parliamone, noi ci siamo e siamo disponibili come sempre, ma facciamo una cosa seria.

importanti quantità di denaro, mai viste prima, che devono essere utilizzate in breve tempo, nel modo ottimale.

bisogna semplificare, bisogna fare norme più chiare possibili, perché altrimenti non si parte. Sottolineo anche un altro importante: per i lavori di adeguamento degli edifici scolastici ci sono grandissime difficoltà per il prossimo anno, perché tantissime aziende, vincitrici del bando, si sono tirate indietro, perché non possono più fare i lavori, visto il rincaro delle materie prime. È un problema o no? Vogliamo pensarci seriamente? Quindi, c'è da fare tanto e la Lega è sempre costruttiva e disposta al dialogo, come penso sia stato dimostrato in tutti i modi, ma ci deve essere anche

sicurezza non solo di avere più lavoro, ma di avere più sicurezza sul lavoro. Anche ieri una donna di quarant'anni è morta

quei provvedimenti che pensiamo vadano migliorati per il bene del nostro Paese, dei cittadini e per rispetto soprattutto di chi, purtroppo, a causa della pandemia ha perso il lavoro, ha perso la propria attività, ma soprattutto ha perso i propri cari e ha visto la propria vita distrutta. Dobbiamo ridare speranza a chi e a chi non ha più trovato un futuro nell'immediato. Dobbiamo ridare un futuro alle persone, perché ne abbiamo la piena responsabilità

È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà. oggi in quest'Aula stiamo discutendo due tra i provvedimenti più importanti della nostra attività istituzionale: il rendiconto di gestione per l'anno 2020 e l'assestamento al bilancio dello Stato per l'anno 2021. Con il Rendiconto generale dello Stato il Governo comunica a noi parlamentari il risultato della gestione finanziaria dell'anno appena concluso, mentre con l'assestamento vengono simultaneamente aggiornate le previsioni riportate nell'ultimo bilancio approvato e si avviano i lavori per la prossima legge di bilancio. Noi tutti dovremmo dedicare molta attenzione a questi due provvedimenti, analizzandone ogni singola voce per comprendere meglio come sta funzionando lo Stato, qual è l'impatto delle nostre scelte politiche e dov'è necessario intervenire per correggere le disfunzioni. Purtroppo questo non accade e si perde una grande occasione, quella della consapevolezza, lo strumento più importante che abbiamo a disposizione e che ci aiuterebbe a trovare le soluzioni per risolvere i problemi. Il Parlamento è sempre più attratto dalla legge di bilancio, ma perde di vista le grandi informazioni che arrivano oggi in quest'Aula attraverso l'intervento dei due relatori e gli interventi che stiamo facendo per spiegare cosa appunto sta accadendo allo Stato. L'analisi finanziaria riportata in questo rendiconto riguarda un anno straordinario, il 2020, l'anno nel quale la pandemia da Covid-19 ha fatto sentire tutti i suoi effetti negativi, mettendo a dura prova lo Stato ed i cittadini. Infatti, i valori economici finanziari e patrimoniali in esso riportati misurano il disagio cui è stato sottoposto il nostro Paese, che ha coinvolto tutti gli aspetti della nostra vita. Leggendo il rendiconto relativo agli anni precedenti, emergeva che venivamo già da una situazione finanziaria che presentava diverse criticità. Ad esempio, sollecitati dall'Europa al rispetto del Patto di stabilità abbiamo sempre dovuto prestare molta attenzione alla situazione del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, il PIL, un indice molto conosciuto da quasi tutti i cittadini. Non siamo, però, riusciti a mettere in atto quei provvedimenti e le riforme attesi da anni, necessari per migliorare i valori di questo indice. In fondo, sarebbe stato semplice: bastava far crescere il prodotto interno lordo, prestando attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. In alternativa, si potevano attuare misure per ridurre il debito pubblico oppure conseguire entrambi i risultati. Tutto ciò, però, non è stato fatto. Poi è scoppiata la pandemia da Covid-19, che ha fatto emergere tutte le debolezze del nostro Paese, a partire dalla gestione del sistema sanitario pubblico, che ha mostrato tutta la sua fragilità rispetto ad uno dei fenomeni più prevedibili a livello mondiale: il contagio da virus. Lo stesso rapporto Stato-Regioni è stato messo a dura prova proprio sulla gestione della sanità, la materia concorrente simmetrica per eccellenza, trasferita alle Regioni in funzione della riforma del Titolo V della Costituzione. Anche su questo tema, che riguarda il corretto funzionamento della pubblica amministrazione a livello centrale e periferico c'è molto su cui riflettere. In pratica, abbiamo avuto la riprova che una determinata modalità di organizzare la non ha dato il meglio di sé; questo rispetto, ad esempio, al tema delle autonomie, che va attenzionato facendo tesoro dell'esperienza avuta nell'ambito sanitario. La pandemia ha anche condizionato e limitato i rapporti sociali, creando dei forti disagi al sistema economico, generando una crisi della domanda. Ciò ha avuto ripercussioni sulle attività imprenditoriali e su quelle professionali, interessando quasi tutte le categorie lavorative. È stata limitata la possibilità per gli studenti di frequentare in presenza le scuole di ogni ordine e grado e per i cittadini di poter interagire agevolmente con le istituzioni. A fronte di quanto appena riportato sul 2020, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 abbiamo dovuto adottare misure straordinarie, che hanno avuto un forte impatto sul bilancio dello Stato, sia per quanto riguarda le risorse stanziate, ma anche per quanto riguarda l'andamento della gestione e la realizzazione della spesa. Porto alcuni esempi. Con il decreto cura Italia abbiamo adottato misure per potenziare il Servizio sanitario nazionale e dare sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese più colpite dalla crisi; con il decreto liquidità abbiamo adottato, fra le altre, misure per facilitare l'accesso al credito e gli adempimenti fiscali per le imprese; con il decreto rilancio abbiamo adottato misure in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali. Con il decreto Covid-19 agosto abbiamo adottato ulteriori misure per il sostegno ed il rilancio dell'economia; con i decreti ristori abbiamo integrato in un solo disegno di legge ben quattro provvedimenti in materia di tutela della salute, di sostegno ai lavoratori e alle imprese, di giustizia e sicurezza. Nel complesso, questi provvedimenti del 2020 hanno immesso nel bilancio dello Stato risorse aggiuntive per oltre 205 miliardi di euro, con il Parlamento impegnato a votare gli scostamenti di bilancio per garantire la copertura finanziaria in virtù della sospensione temporanea dei vincoli del Patto di stabilità. Inoltre, è doveroso da parte mia, visti i precedenti interventi, ricordare la grande funzione sociale assolta dal reddito di cittadinanza, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle già dal 2019. cittadinanza è il più potente strumento di sostegno ai soggetti svantaggiati, che ha consentito la sopravvivenza di milioni di persone e la tenuta del Paese in un momento di grande crisi sociale. E lo state dimenticando! In sintesi, in piena crisi Covid, il Governo a guida del presidente Conte e il Parlamento hanno lavorato costantemente per potenziare il Sistema sanitario nazionale, per sostenere le imprese, per aiutare i lavoratori autonomi e dipendenti e per supportare il sistema scolastico e quello giudiziario. Tutto ciò ha determinato un inevitabile peggioramento delle voci che compongono il Rendiconto generale dello Stato. Senza entrare nel dettaglio degli importi, si può affermare che sono diminuite le entrate e che sono aumentate considerevolmente le spese. Dall'esame della gestione patrimoniale 2020 emerge un'eccedenza passiva di 2.215 miliardi di euro, con un peggioramento di quasi 300 miliardi di euro rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019. Questo risultato ha un carattere straordinario, in quanto non rispecchia il *trend* rilevato negli ultimi anni. Per quanto invece riguarda l'assestamento per l'anno 2021, le variazioni proposte con il disegno di legge evidenziano un peggioramento del saldo netto da finanziare, che corrisponde alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si assesta su un valore di meno 232,8 miliardi, rispetto a una previsione iniziale di meno 193,5 miliardi, con un peggioramento di circa 40 miliardi dovuto alle variazioni apportate per la necessità di adottare altri provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza da Covid-19, per la quale in Parlamento abbiamo autorizzato il ricorso a un ulteriore indebitamento. A un bilancio dello Stato che in fase di rendicontazione e di assestamento evidenzia delle criticità così importanti, condizionate da una pregressa situazione già negativa e aggravate da motivazioni di natura sanitaria, per rilanciare il nostro Paese, tutelare gli interessi dei cittadini, salvaguardare e valorizzare il territorio e l'ambiente, possiamo rispondere in un solo modo: eseguire concretamente nei tempi prestabiliti il PNRR. Le risorse finanziarie concesse all'Italia dall'Unione europea, grazie soprattutto all'impegno del Governo Conte *(Applausi)*, che, abbinate a quelle previste con il Fondo di solidarietà e coesione, ammontano a circa 237 miliardi di euro, rappresentano l'opportunità per rendere il nostro Paese moderno e competitivo, sia in ambito europeo che mondiale. L'Unione europea ha concesso queste risorse indicando tra le priorità quella di colmare il divario di sviluppo economico e sociale tra Nord e Sud Italia. Mi preme sottolineare che per il Nord è necessario avere un Sud più sviluppato, che possa concorrere insieme al Nord per rendere l'Italia una Nazione solida e un punto di riferimento forte nel sistema economico mondiale. Le riforme che adotteremo a supporto del PNRR dovranno andare in questa direzione. La riforma della giustizia, del fisco, della pubblica amministrazione e del mercato del lavoro sono passaggi propedeutici fondamentali per assicurare i risultati attesi dal PNRR; non ci sono alternative. Il MoVimento 5 Stelle ha finora dimostrato un grande senso di responsabilità verso il Paese, garantendo il sostegno al Governo anche quando i provvedimenti adottati non erano totalmente in linea con i propri valori portanti (vediamo l'ultima riforma della giustizia in ambito penale). Ma siamo consapevoli dell'eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo, che non riguarda solo l'Italia. Abbiamo un tempo limitato per far sì che il nostro Paese riparta senza perdere questa opportunità di rilancio, che vede necessariamente prevalere la collaborazione e la coesione a tutti i livelli. Per queste ragioni, credendo nella validità del PNRR, annunzio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sui disegni di legge Rendiconto di gestione 2020 e assestamento 2021.

vorrei rendere noto all'Assemblea che, da notizie di stampa, pare sia in corso un consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, all'interno del quale sembra essere stato proposto, dal ministro Giovannini, il nome di Ugo de Carolis, ex amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ex uomo di Benetton e uomo di Castellucci, amministratore delegato di Atlantia.

una nomina che va contro i genovesi, le vittime del ponte Morandi e i loro familiari.

parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge recante: «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2021, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021. Infine, il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 1), l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (articolo 2), modifiche e integrazioni ai compiti dell'Osservatorio sullo spettacolo (articolo 3) e l'attivazione a carico dell'INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 4), appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono altresì conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.»

vigente. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16 con la discussione delle risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite affari esteri e difesa sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. *(La seduta, sospesa

sulle presunte voci inerenti alla nomina di Ugo de Carolis come amministratore delegato di ANAS. Tutti sappiamo - lo ha ricordato anche il collega che è intervenuto questa mattina che Ugo de Carolis è uomo vicino ai Benetton e all'amministratore delegato Castellucci. È conosciuto per essere stato amministratore delegato di Aeroporti di Roma

una storia che mai più avremmo voluto vivere e ripetere. *(Applausi)*. Io chiedo - com'è stato fatto anche da altri anche alla Camera dei deputati - che il ministro Giovannini intervenga direttamente e urgentemente

che vanno oltre la parte concreta della nomina, nascondono un magone, perché una cosa del genere mai ce la saremmo aspettata da un Governo e da un Ministro. è difficile per me pronunciare queste parole trattenendo una rabbia che - spero - sia inerente soltanto a un tentato affronto e non a una realtà, sulla quale crediamo di fare una forte retromarcia.

mi associo alle parole che ho sentito ora dal collega Bruzzone. Siamo a pochi giorni dal 14 agosto. Credo che non solo per nessun genovese, ma per nessuna persona in Italia e forse nel mondo sia possibile dimenticare il crollo del ponte Morandi, la tragedia

c'è una questione legata alla ferita della città. C'è un processo in corso ed è evidente comunque che ci sono state responsabilità.

non si facciano nomine che possano offendere la città di Genova, le vittime e siano un dimenticare quanto avvenuto. Voglio dunque che arrivi forte e chiara anche la voce del Partito Democratico su questa vicenda.

di miliardi, nonostante fossero i responsabili del fatto di non aver effettuato le manutenzioni sul ponte Morandi. Ora si vuole anche nominare come presidente dell'ANAS un uomo a loro legato, legato all'ex amministratore di Atlantia Castellucci? È questo che si vuole? Com'è possibile che i colleghi che hanno parlato non dicano ai loro partiti che questo non deve essere consentito al Governo? Non potete dare la fiducia al Governo e poi consentire uno scempio

grazie a tutte

un intervento del senatore Toninelli. Non avrei mai pensato di farlo in tutta questa legislatura, e dico la verità.

anche perché fra poco è l'anniversario del crollo del ponte Morandi, in una logica che a questo punto sembra una sorta di *fil rouge*. E mi mi viene da sorridere che una parte della maggioranza abbia aderito a certe scelte. fucilare, disintegrare e cancellare quel pezzo di società, la gestione Benetton, Atlantia e compagnia bella; poi, gli abbiamo comprato, con 9,5 miliardi di euro degli italiani, le azioni e siamo diventati proprietari del 90 per

ci fa particolarmente specie che un atteggiamento del genere si ripeta e che il Governo non si sia sentito nemmeno responsabile di convocare la maggioranza per dare un'indicazione rispetto a ciò. attuale non è un Governo scollegato dal sistema parlamentare: è il Parlamento che dà l'indirizzo; è bene che non ce lo dimentichiamo mai. E su tale questione ritengo che non possiamo assolutamente indietreggiare. Spero che questo corale disappunto di inopportunità si trasformi in un altolà alla scelta fatta.

dovrebbe diventare, nonostante i suoi trascorsi opachi, non brillanti, molto discutibili, il nuovo amministratore delegato di ANAS all'interno dell'accordo tra ANAS e Ferrovie.

Eppure, colleghi della maggioranza, non basta - scusate il termine - ululare alla luna. Se siete veramente convinti che la scelta è sbagliata; se siete convinti, come ha appena detto il senatore Mallegni, che il Parlamento deve esercitare il proprio ruolo fino in fondo e fare sentire la sua voce, c'è un modo per trasformare

completare l'*iter* autorizzativo della nomina del signore in questione. Questo è un modo per esercitare la sovranità del Parlamento. Tutte le altre sono belle discussioni che lasciano il tempo che trovano.

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,

Signor Presidente, con questa deliberazione oggi il Senato è chiamato all'esame del provvedimento di autorizzazione alla partecipazione alle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga, come dal contenuto delle risoluzioni in esame, con la procedura introdotta dalla legge n. 145 del 2016. Si tratta di due risoluzioni sulle nuove missioni che sono state introdotte nel 2021. Per quanto riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo interverrà il senatore Vescovi, che con me ha partecipato alla redazione delle risoluzioni. La deliberazione delle missioni, approvata con le risoluzioni oggetto del presente dibattito dalle Commissioni riunite 3a e 4a, si inserisce in uno scenario di sicurezza reso più complesso e instabile dalla pandemia. La fase storica che si sta aprendo ha moltissime incognite, come emerso in tutte le audizioni svolte durante l'*iter* di questo provvedimento. Il rischio molto concreto è che la pandemia accentui le dinamiche di frammentazione e maggiore conflittualità che lo scenario geopolitico già mostrava chiaramente da diversi anni. In particolare, è ancora da esplorare quale sarà l'impatto sui Paesi fragili, con Governi e istituzioni deboli, con condizioni sociali critiche, con conflitti in corso e con sistemi sanitari deboli o inesistenti. Basti pensare a come, analogamente al resto del mondo, il coronavirus abbia portato a una sospensione della maggior parte delle attività economiche e commerciali nel Maghreb, per esempio. Paesi che avevano il turismo e gli investimenti stranieri al centro delle proprie economie hanno visto questi settori azzerati in un contesto già caratterizzato da numerose vulnerabilità. Ed è alquanto dubbia la capacità dei Governi locali di dare una risposta a istanze e rivendicazioni di carattere socio-economico e politico e di proseguire un percorso di democratizzazione. Ne è la prova la crisi di questi giorni in Tunisia, ma anche le agitazioni in Marocco e in Algeria. Il senso del provvedimento di oggi sta nell'assegnare alle Nazioni più avanzate del pianeta, ancora di più che nel passato, il compito di operare congiuntamente, al fine di gestire le instabilità e continuare a sostenere il sistema di *governance* che ha come riferimento l'ONU e il diritto internazionale. Le linee di azione dell'Italia si fondano su principi base che orientano e sovrintendono alla nostra politica estera di sicurezza; principi che seguiamo da molti anni e che discendono dal secondo periodo dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Mi riferisco alla nostra adesione al sistema di relazioni e istituzioni basato sulle Nazioni Unite e sulle altre organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale e, quindi, alla nostra scelta per una gestione multilaterale delle crisi e per conferire stabilità, continuità, capacità e programmazione all'azione della comunità internazionale a favore della stabilità e dello sviluppo pacifico. Le missioni internazionali rappresentano un'assunzione di responsabilità per un Paese come il nostro, che si è sempre schierato dalla parte della tutela del diritto internazionale e vanta un impegno di lunghissimo periodo a favore dei diritti umani, per la gestione multilaterale delle crisi e per il rafforzamento delle organizzazioni multilaterali, in uno scenario mondiale sempre più esposto a rischi di conflitto. Tra l'altro, possiamo ben dire che, se vogliamo essere fruitori di sicurezza nell'interesse del nostro Paese, dobbiamo con coraggio e responsabilità contemporaneamente essere produttori di sicurezza. il contributo dell'Italia è quello della partecipazione ad oltre 40 missioni, con una presenza media di circa 6.500 unità di personale, con un massimo autorizzato di circa 9.500, con un *focus* specifico come indicato dal ministro Guerini in sede di audizione - sul Mediterraneo allargato, che rappresenta una priorità assoluta per il nostro Paese. La faglia identitaria e confessionale che sta attraversando la Penisola arabica favorisce dinamiche di riposizionamento dei principali attori regionali e globali, con possibili ricadute sugli interessi industriali ed energetici nazionali. La rimodulazione dell'impegno statunitense (in Afghanistan, in Iraq e in Siria, ad esempio) e l'attivismo di Turchia e Russia hanno determinato nuovi squilibri che potrebbero essere origine di ulteriori crisi. A proposito di Afghanistan - come viene sottolineato nella risoluzione di proroga - nonostante la conclusione della missione Resolute support, si ritiene che l'Italia debba mantenere una presenza forte nell'ambito di uno sforzo comune della comunità internazionale per garantire il mantenimento dei progressi, in particolar modo con riguardo alla condizione femminile, realizzati finora anche grazie a un impegno gravoso da parte di tanti Paesi dal punto di vista delle perdite di vite umane, prima ancora che dal punto di vista finanziario. Nel Sahel e nel Corno d'Africa l'instabilità politica e le fragilità delle istituzioni statuali costituiscono una fonte di criticità per l'Italia in termini di sicurezza e di possibile avvio di nuovi flussi migratori. Nei Balcani ancora si assiste a una crescente presenza di diversi attori extraeuropei, con pesanti ricadute in termini di influenza politica, ma anche di flussi migratori. A fronte di tali scenari, l'Italia continua a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in atto in Libia. Credo sia utile ragionare sul motivo della nostra presenza in Libia e avere una visuale completa. L'impegno dell'Italia verso quel Paese, in atto da molti anni, si è sempre svolto in ambito ONU e a favore di un maggior ruolo dell'Unione europea. Abbiamo inteso svolgere per ovvie ragioni un ruolo di primo piano, ma sempre coordinato e con lo sguardo rivolto alle organizzazioni multilaterali che sono il nostro punto di riferimento. Questo sulla base di un presupposto evidente: credo non ci siano dubbi che quella per la stabilizzazione della Libia sia una questione di rilevanza assoluta per le conseguenze sull'equilibrio e la sicurezza del Nord Africa e dell'intero Mediterraneo; questo per l'Unione europea, ma soprattutto per l'Italia. La Libia ha bisogno del massimo sforzo possibile dell'Italia e della comunità internazionale per scongiurare il rischio di una destabilizzazione che sarebbe un disastro; uno sforzo che, per avere successo, non può non essere coordinato e vedere un maggior ruolo dei Paesi dell'Unione europea (su questo interveniamo anche nella risoluzione). Ma, per avere questo risultato, non possiamo non essere noi, per posizione, storia, legami e cultura, ad avere un ruolo speciale. Ci troviamo nel mezzo. Da anni svolgiamo un ruolo speciale senza essere riusciti a raggiungere un più decisivo impegno comune europeo. Il punto è che un nostro arretramento renderebbe la situazione è ancora più difficile. Per essere chiari e per non essere fraintesi, se la cooperazione è indispensabile, non ci sono dubbi che debba basarsi su alcune condizioni in merito ai diritti umani e alla tutela dei più vulnerabili, ma occorre anche essere chiari su altri punti. Le missioni di cooperazione nel loro complesso, comprese quelle bilaterali e tutte quelle su cui interveniamo in Libia, sono inserite nel più ampio impegno politico dell'Italia per contribuire attivamente alla stabilizzazione e pacificazione, senza le quali ben pochi passi potrebbero essere fatti in tema di protezione e diritti umani. La nostra azione in Libia è storicamente e fattualmente indirizzata a favorire un più ampio coinvolgimento della comunità internazionale e, in particolare, dell'Unione europea. Ed è sicuramente necessario operare per garantire in Libia e nei centri di detenzione la possibilità di accesso e di azione alle organizzazioni internazionali che operano nel campo dell'immigrazione e dell'assistenza umanitaria. Con queste premesse, nella risoluzione

a verificare le condizioni per il superamento della missione di assistenza alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi - di cui alla scheda trasferendone le funzioni ad altre missioni, con l'obiettivo, appunto, di consolidare il ruolo dell'Italia in Libia e potenziare il coinvolgimento europeo. Questo per sottolineare come la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia non solo non solo un elemento fondamentale della nostra politica estera di difesa, ma anche uno dei nostri tratti identitari nel quadro di relazioni bilaterali, di adesione a trattati, accordi e legami che caratterizzano la nostra collocazione e le nostre priorità nel contesto internazionale. Concludo formulando un ringraziamento alle nostre Forze armate per l'impegno dimostrato, con serietà e professionalità riconosciuta a tutti i livelli, ribadendo ancora una volta che il nostro Paese vanta un impegno di lungo periodo, rimanendo tra i più importanti Paesi contributori, sia in termini di personale impiegato sia per quanto concerne il contributo finanziario. Le Commissioni affari esteri e difesa riunite hanno valutato favorevolmente i contenuti della deliberazione del Consiglio dei ministri. Sono state accolte alcune istanze emerse nel corso del dibattito, alcune già evidenziate. In un'altra viene rilevata l'esigenza di verificare una maggiore semplificazione del procedimento di autorizzazione parlamentare per l'avvio e la proroga delle missioni internazionali, ritenendo - come ribadito nella risoluzione - che, anche a seguito delle criticità emerse durante i primi anni di applicazione della legge quadro, sarebbe opportuno valutarne un intervento di adeguamento. Con quanto premesso, le Commissioni riunite propongono all'Assemblea di autorizzare le missioni e le attività di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri nei termini previsti dalle risoluzioni

Signor Presidente, per quanto mi riguarda, vorrei illustrare le nuove sei missioni con partecipazione italiana: la partecipazione di personale militare alla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia; l'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per l'attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz; il riconoscimento, quale operazione finalizzata a eccezionali interventi umanitari, dell'operazione definita Emergenza cedri in Libano;

a questa relazione. Io sono convinto che la grandezza di un Paese venga misurata dalla politica estera. Per questo, mi permetto di ringraziare il presidente Draghi, che, con la sua autorevolezza, in diverse occasioni ha dimostrato un netto cambio di passo, in particolar modo nello scenario libico e nel chiarire i nostri rapporti con la Turchia, oltre aver cristallizzato, fuori da qualsiasi ambiguità, la nostra appartenenza all'Alleanza atlantica e ai valori del mondo occidentale.

Ricordo che eventuali ordini del giorno al testo delle risoluzioni approvate dalle Commissioni riunite 3a e 4a potranno essere presentati entro la conclusione della discussione congiunta.

dirò no con il mio voto ai finanziamenti per le milizie libiche, perché tutti noi sappiamo tutti noi sappiamo che i gruppi delle milizie libiche, confederati nella cosiddetta "guardia costiera libica", sono gli stessi signori della guerra che sfruttano il traffico di esseri umani e che gestiscono i campi di detenzione. Sono milizie accusate di crimini contro l'umanità, per aver violato e per continuare a violare migliaia di vite di migranti e di richiedenti asilo, ridotti in schiavitù per evitare che arrivino sulle nostre coste. E questa ecatombe nel Mediterraneo, a poche miglia da noi, è il simbolo del fallimento morale e politico delle democrazie europee, della cecità e del cinismo delle classi dirigenti. I campi dell'orrore in Libia sono un buco nero nella storia dell'umanità e per essi verremo giudicati dalla storia, politicamente prima ancora che moralmente, perché nessuno può più dire di non sapere quello che avviene nei campi libici. Lo sappiamo, perché ripetutamente, ormai da anni, lo dicono le denunce dell'ONU e del Consiglio d'Europa, lo dicono gli atti della procura internazionale dell'Aja, lo dicono le foto e i filmati delle inchieste, tra cui quelle coraggiose dei giornalisti italiani, che non finiremo mai di ringraziare per il loro impegno civile. Lo dicono le testimonianze dei sopravvissuti, la voce straziante delle donne torturate e violentate, degli uomini sequestrati e lasciati morire, delle bambine e dei bambini incatenati, percossi, seviziati, che numerosi tentano il tentano il suicidio per disperazione e per fame. Non c'è giustificazione a tutto questo, non può esserci giustificazione a tutto questo. Non c'è alta politica che tenga, non c'è malinteso realismo politico, non c'è ragione di Stato che possa renderci conniventi con tutto questo. Eppure, Presidente, quei campi sono legittimati e contemplati da un accordo sottoscritto tra Italia e Libia; e questo è inaccettabile. Un accordo tra due Governi, mai passato in Parlamento; e questo è inaccettabile. Un accordo che non è mai stato riscritto, nonostante gli impegni presi anche in quest'Aula. È sulla base di quel *memorandum* che esiste un'area cosiddetta di "ricerca e soccorso" libica nel Mediterraneo. Nonostante la Libia non abbia mai sottoscritto le convenzioni internazionali sul rispetto dei migranti, noi deleghiamo loro a intervenire al nostro posto, a respingere al nostro posto, a catturare e rinchiudere nei campi, perché questo fanno le milizie libiche che noi sosteniamo. Altro che soccorso, Presidente. C'è un video di pochi giorni fa, nel quale una motovedetta libica, donata dall'Italia, viene ripresa mentre spara su un barcone carico di persone, tentando di speronarlo. Questo avviene e questo continua ad avvenire. Per questo, Presidente, voterò no. Per questo, insieme al senatore Nannicini e al senatore D'Arienzo, pronunciamo il nostro no in quest'Aula e di fronte all'opinione pubblica, perché nulla è cambiato, a dispetto dell'ipocrisia e delle promesse. La situazione, anzi, nell'ultimo anno è peggiorata. "Medici senza frontiere", uno degli ultimi baluardi rimasti, ha sospeso le attività nei centri, denunciando l'aumento esponenziale delle violenze negli ultimi mesi.

guerra civile e agli interessi della Turchia, della Russia o di altri. C'è un altro modo per stare in Libia e per stare con la Libia

va interrotta questa missione, che ha rafforzato il sistema dei campi di tortura, anziché smantellarlo. Va scritto un nuovo accordo - lo chiediamo con forza - che coinvolga Europa, Africa, Nazioni Unite, organizzazioni umanitarie, organizzazioni non governative e società civile e che affronti le cause strutturali di un fenomeno migratorio che è epocale e che coinvolge milioni di persone, che fuggono da atrocità indicibili e che nessun muro

perché solo così l'Italia e l'Europa potranno riscattare il proprio ruolo e la propria funzione storica e svolgere una *leadership* che sia credibile, vera e riconosciuta, nel Mediterraneo e nel mondo. *(Applausi)*.

ha ben ragione il relatore quando dice che le missioni internazionali a cui l'Italia partecipa sono uno strumento importante della proiezione italiana sul fronte internazionale. Esse rappresentano spesso la faccia dell'Italia anche nei luoghi più disperati e i nostri militari, a cui va tutto il nostro ringraziamento, sono apprezzati da tutti per la loro capacità professionale, ma anche per l'umanità che mettono nelle varie missioni, normalmente al fianco dei più fragili, dei più deboli e in operazioni e in opere civili.

necessario valutare bene, missione per missione, senza automatismi, ma considerando i risultati raggiunti e il contesto generale che, almeno nel Mediterraneo, è in rapidissimo cambiamento. Signor relatore, lei ha parlato di Mediterraneo allargato: è vero, ma questo Mediterraneo allargato è tutto in subbuglio. Intanto le preannuncio

C'è poi la Libia - di cui avete parlato e su cui tornerò - ma recentemente abbiamo avuto anche l'esplosione della Tunisia, attualmente in una tregua instabile e altrettanto poi il Marocco, con la questione di Ceuta e Melilla e altre questioni bilaterali aperte con la Spagna. Insisto a dire che esiste poi un buco nero di cui poco ci occupiamo - forse perché poco ce ne possiamo occupare - che è l'Algeria.

Le Nazioni Unite già ci parlano di 30.000 persone in marcia per la fuga. Ma voglio almeno essere sicura che tutti coloro che hanno

perché non è una missione internazionale. La scheda n. 48 riguarda la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Si tratta di un accordo bilaterale abbastanza, se non del tutto, sconosciuto.

persone e di diminuire i salvataggi in mare, che non facilitiamo di sicuro, dobbiamo spezzare qualunque connivenza a terra sul territorio libico.

È veramente inaccettabile dal mio punto di vista - ma è bene che questa discussione avvenga al Senato - che ci si assuma la responsabilità di mandare indietro nei carceri - si fa per dire - per essere torturati, disperati migranti che cercavano solo una vita migliore.

Va ripensato in particolare il nostro impegno bilaterale con la Libia, che dura dall'accordo di partenariato a cui già mi opposi. È vero opposi. È vero che per ora molti Stati europei sono sordi, ma proprio per questo dobbiamo insistere e prepararci ai nuovi arrivi.

Non dobbiamo ergerci a giudici dei diritti umani o dare lezioni ad altri, perché anche noi non andiamo fortissimo.

Anche noi avremmo un gran bel lavoro da fare nel nostro Paese per un'immigrazione rigorosa e nello stesso tempo umana, quindi non ci ergiamo a maestri dei diritti umani, perché non lo siamo; non lo siamo; tuttavia, proprio perché ne abbiamo esperienza, dobbiamo assolutamente insistere perché questo sia il cammino di marcia verso cui tendere. In questo quadro la Libia non c'è, non ci sta

a cosa è servita questa cooperazione con la Libia. È servita a portare indietro e a far torturare delle persone, certamente non ha contribuito a stabilizzare il Governo del Paese. questo debba saperlo chiunque si assuma altre responsabilità, ma io penso sia più serio sospendere questa missione e ripensare complessivamente a come vogliamo porci

Signor Presidente, le missioni internazionali sono un aspetto importantissimo per le nostre Forze armate e per la nostra politica estera in generale. L'Italia è il secondo contributore in termini di truppe alle missioni internazionali della NATO, ha avuto delle posizioni di vertice e presto ne avrà un'altra molto importante di cui parlerò fra poco. È un orgoglio ed è motivo di prestigio e naturalmente per questo va soprattutto la riconoscenza agli uomini e alle donne delle Forze armate che partecipano con grandissima capacità e con straordinari risultati a queste missioni, riscontrando l'apprezzamento non soltanto nostro, del Governo e dell'opinione pubblica italiana, ma dei comandi degli altri Paesi che spesso giudizi estremamente positivi sulle nostre truppe, sulla loro preparazione, ad esempio sulla particolarità dei Carabinieri, che hanno sia una preparazione di forza di polizia, sia uno

grazie a tutte

una volta semplicemente per citare l'iniziativa del *Mediterranean* *dialogue* (il dialogo mediterraneo) e l'altra per ricordare che esiste l'*hub* di Napoli di Napoli volto verso il Mediterraneo. In sostanza, il Mediterraneo è completamente ignorato. C'è tutto un versante europeo

continuerà a essere il secondo contributore in termini di truppe e un italiano sarà a capo della delicatissima missione in Iraq.

del Nord Africa e dell'Africa subsahariana) abbia la sua influenza. Si tratta di cose che ci toccano tutti i giorni. Si parla dell'arrivo degli immigrati, che è una realtà quotidiana. Comunque la si veda, è un aspetto importantissimo. Da dove arrivano gli immigrati e da cosa sono spinti? Sono spinti dagli squilibri presenti nel Mediterraneo e dai problemi nel Nord Africa e anche nell'area sahariana e subsahariana. Dunque, non è possibile

Spetta al Governo far pesare il ruolo dell'Italia. In questo ambito possiamo e dobbiamo far pesare il nostro impegno nelle missioni internazionali e, se vogliamo farlo pesare all'estero, dobbiamo mostrare di averne grande considerazione in Italia.

È vero, il Ministro della difesa è andato a Herat e ha partecipato alla cerimonia, ma francamente è difficile pensare che questo tocchi l'opinione pubblica italiana.

che si deve alle migliaia e migliaia di uomini e donne che hanno partecipato a questa missione, ai 53 caduti e ai tanti feriti. Cominciamo ad avere considerazione di noi stessi in Italia e facciamola valere

il professor Luigi Manconi, senatore della passata legislatura, si è interrogato sulla soglia oltre la quale non è più possibile proseguire i rapporti con un Paese senza democrazia e senza Stato di diritto dove vengono quotidianamente violati i più elementari diritti umani. Manconi sa che quella soglia si può trovare solo nel rapporto tra la gravità dei fatti e gli obiettivi della missione. Se si cercano la pace e lo Stato di diritto, solo una saggia e lungimirante valutazione politica può discernere tra le conseguenze di una rottura e l'utilizzo degli strumenti della diplomazia. Dopo il 1989, finito l'equilibrio nucleare tra USA e URSS, il mondo ha sbandato ed ancora non si è ripreso, ed oggi l'unico equilibrio possibile è quello molto difficile e instabile di un multilateralismo attento e pragmatico. Da questo assunto nascono le missioni internazionali, che preservano quell'ordine mondiale che da decenni tiene il mondo in precario equilibrio. Oggi l'Italia opera in cinquantanove missioni, cercando di contribuire a garantire pace e stabilità in Paesi dove frequentemente - sottolineo «frequentemente» non ci sono né democrazia né Stato di diritto né rispetto per i diritti umani. Ed è su queste missioni che dobbiamo interrogarci. Qual è la soglia oltre la quale l'Italia deve sentire il dovere di andarsene e lasciare quei Paesi al loro destino? Oppure, se decide di restare, che tipo di assistenza può essere data senza venir meno ai doveri imposti dalla nostra democrazia? Davanti a tante conclamate atrocità, di cui hanno parlato i colleghi Verducci e Bonino, l'Italia per moralità politica dovrebbe interrompere il suo lavoro di addestramento della Guardia costiera libica. Ma siamo certi che così facendo non si spezzerebbe quel tenue filo che ancora collega i regimi libici e la democrazia italiana? Siamo certi che così non si aggraverebbero irrimediabilmente le condizioni di chi oggi in Libia vive in balia della violenza? Devo dire che io questa certezza non ce l'ho. Davanti a questo dilemma penso che dobbiamo apprezzare la decisione delle Commissioni del Senato che impegnano l'Italia a coinvolgere l'Europa nell'addestramento, a partire dal prossimo anno, della Guardia costiera libica, così superando la dimensione nazionale della nostra missione.

Le condizioni della Libia sono vitali per l'Italia ed era già così ai tempi di Gheddafi, che non ci piaceva ma con il quale tenevamo buoni rapporti. Oggi la stessa Francia si è forse pentita del *raid* che ha destituito il *ràis*. Per cercare di capire, voglio seguire il riferimento di Emma Bonino al ritiro americano e italiano dall'Afghanistan e osservare come, di giorno in giorno, si aggravino i suoi effetti negativi, non solo geopolitici, ma anche sulla libertà e sulla vita di migliaia di afghani. Se oggi Peter Hopkirk dovesse riscrivere il suo splendido romanzo «Il grande gioco» sull'Afghanistan dell'Ottocento, inserirebbe nuovi attori e amplierebbe il teatro dell'azione. le tensioni in Afghanistan venivano da un intreccio insolubile di contrapposizioni storiche: grandi potenze e piccoli potentati, eserciti regolari ed organizzazioni terroristiche, interessi politici, economici e commerciali contrastanti, trame di servizi segreti, guerre dichiarate e guerre sporche, traffici di droga, tradimenti, doppio gioco e lotte di religione. Questa era ed è tuttora la realtà, non solo dell'Asia centrale, ma anche della diversissima Libia. Parliamo di Paesi che hanno storie antiche alle spalle e di cui la comunità internazionale, Italia compresa, deve tenere conto. Da secoli l'Asia centrale, il Medio Oriente, la Costa Sud del Mediterraneo sono al centro di grandi interessi strategici e le tensioni, le guerre, le stragi e gli attentati appaiono così connaturati a vicende storiche antiche da farci dubitare del successo delle missioni internazionali di pace. Ma non possiamo mollare perché sappiamo che, se vogliamo che in quelle regioni torni la pace, dobbiamo favorirne la stabilizzazione politica anche con la nostra presenza. I confini dell'Europa a Est, a Nord e a Sud sono diventati più vulnerabili. Dopo l'attivismo di potenza russo e turco nel Mediterraneo, quel Mediterraneo allargato cui ha fatto cenno Emma Bonino, che cos'altro deve accadere per convincere l'Europa che senza una comune politica estera e di difesa corre gravissimi pericoli? La storia può insegnare molto. L'assenza di coraggio delle democrazie europee nei confronti del nazismo nascente non ha impedito, né la Seconda guerra mondiale, né l'olocausto. Ricordarlo può aiutarci a comprendere quanto sia pericoloso sottovalutare la debolezza della politica estera e di difesa dell'Europa. Le vicende del Medio Oriente, dell'Asia centrale e della Libia chiamano l'Europa non a intervenire in ordine sparso, ma a farlo come un'unica grande nazione che conosce i suoi interessi e i suoi doveri. In Afghanistan gli Stati Uniti avevano 2.500 militari e l'Italia era presente con 895 unità ed eravamo il terzo contingente. Ma, se l'Europa fosse stata uno Stato federale, il suo contingente in Afghanistan sarebbe stato di gran lunga il più numeroso e molto più significativa la sua influenza. Oggi la nostra richiesta di una maggiore presenza dell'Europa in Libia ha un segno europeista, ma, un conto, è voler fare dell'Europa una federazione, un altro è limitarsi a difendere doverosamente i nostri concreti interessi nazionali. L'Europa ci sta procurando i vaccini e dall'Europa vengono gli aiuti alla nostra economia ed è tutto necessario, ma la geopolitica, la Libia, l'Asia centrale e il Medio Oriente ci dicono che serve anche un europeismo di vista più lunga, un europeismo che sappia ambire ad un'Europa federale in grado di esprimere una comune volontà nella gestione, non solo dell'economia, ma anche della politica estera e di difesa. Qualcuno ha detto che raramente i contemporanei riescono a percepire le grandi trasformazioni che avvengono sotto i loro occhi e forse è per questa ragione che l'Europa non riesce a vedere quanto seri siano i rischi che sta correndo. Concludo. Il passaggio da Trump a Biden ha messo fine a un incubo, ma ha anche messo nuovamente in evidenza le debolezze strutturali di un'Europa che non può continuare a pensare che la propria sicurezza rimarrà in eterno affidata alla forza dell'alleato americano. Il disimpegno dall'Afghanistan e le vicende della Libia debbono far maturare l'idea di quanto sia necessaria una vera difesa europea, una difesa che abbia dietro una politica e una forza armata europea. Grazie

Tutto questo, però, lo stiamo facendo ad agosto. Colleghi, ci rendiamo conto che tutto ciò di cui stiamo parlando è già in gran parte è avvenuto e che stiamo ratificando ciò che è già passato da otto mesi?

violare la legge del 2016, fatta appositamente perché il Parlamento potesse valutare approfonditamente le varie missioni cui giustamente partecipa l'Italia per contribuire a mantenere la pace nel mondo; non si può discuterle ad agosto. È un'aberrazione, è un'abdicazione sostanziale al dovere del Parlamento di dare l'indirizzo politico e soprattutto di definire l'interesse nazionale, come in parte stava cominciando a fare nel proprio intervento il senatore Zanda. Per il resto, vorrei richiamarmi preliminarmente all'intervento del collega Verducci, che bene ha rappresentato la situazione in Libia e anche la situazione dei soccorsi, ricordando le immagini che tutti abbiamo visto e nessuno può dire di non sapere, né in questo Parlamento né nell'opinione pubblica. Non esiste un'azione di soccorso della cosiddetta guardia costiera libica. Sapete perché si dice cosiddetta? Perché non esiste una struttura gerarchica unitaria. È composta in parte da miliziani, in parte da ufficiali della Marina

di uomini. Sempre il senatore Zanda si chiedeva fino a che punto lo Stato può trattare con la mafia. Fino al punto in cui non c'è alcun modo per parlare la stessa lingua.

Ci abbiamo perso 53 uomini; il ritorno è stato fatto quasi di nascosto. Bene, a questo punto non possiamo andar via da lì senza proteggere quelle 800 persone e le loro famiglie.

bisogna dar loro il visto per entrare in Italia domani perché dopodomani, uno di loro potrebbe non esserci più. Di cosa parliamo, allora? Di aver fatto il nostro dovere su un pezzo di carta?

semmai possa rispondere subito - quali siano gli impedimenti che ostacolano la messa in sicurezza delle 800 persone, che sono state con noi per tanti anni e hanno protetto gli italiani in Afghanistan. Hanno consentito che gli italiani lavorassero in sicurezza.

noi stiamo finanziando la Guardia costiera libica che è sotto il comando e il controllo dei turchi. Lo sappiamo o non lo sappiamo? Le notizie sono queste: i turchi hanno il controllo di tutti i porti della Tripolitania e nella Tripolitania c'è Tripoli. I porti di Tripoli, da cui partono le due motovedette libiche, sono sotto il controllo turco. Ora noi stiamo finanziando i libici, ma i turchi, in realtà, li manovrano. Il comando e il controllo, fino al 2 luglio 2020, era nostro; lo ha detto il ministro Guerini. Il 7 luglio,

e gli strumenti di comunicazione di questa erano nella disponibilità immediata della cosiddetta Guardia costiera libica. Ma chi c'era della Guardia costiera libica? Un ufficiale di collegamento, il quale andava a bordo, firmava un pezzo di carta («Messaggio di assunzione di responsabilità di coordinamento») e la sua attività finiva. A quel punto, su quella nave - questo è provato - arrivavano le disposizioni di coordinamento, cioè posizione (latitudine e longitudine), unità (quante persone c'erano a bordo)

Queste intercettazioni dimostrano che i libici non sono così cattivi come noi li dipingiamo, perché loro sono dei meri, bassi esecutori. Al comando di chi effettuavano i respingimenti in mare? Nostro: Capitaneria di porto, Guardia costiera,

dall'Italia, da Malta e da Frontex? Allora, i mandanti di quei crimini che sono i respingimenti illegali non sono i libici, siamo noi. noi. Noi oggi dobbiamo dire: basta. Creiamo una discontinuità con questa situazione aberrante, perché la storia ci chiamerà a rispondere; vi e ci chiamerà tutti a rispondere. Nessuno potrà dire: io non ho visto, non sapevo.

di contributo. È però successo che la Presidenza, composta dalla senatrice Pinotti e dal Presidente della Commissione affari

le firme necessarie, ossia un terzo dei componenti la Commissione, le risoluzioni (e lì non si parla più, come nel comma 2, di quelle approvate) vengono in Aula. In questo modo, non facendo venire in Aula le risoluzioni, si conculca il diritto e dovere del singolo parlamentare di valutare la situazione nella sua interezza e soprattutto si limita il voto dell'Assemblea. Attenzione, cari colleghi, voi oggi dovete votare ciò che è già stato approvato; non potete valutare e discutere... Le avevo già dato del tempo supplementare per poter spiegare questo punto di vista, però la prego di concludere.

Approfitto della spiegazione che devo dare al senatore De Falco. È vietato fotografare.

Sapete che non è possibile, quindi vi chiedo di lasciare i banchi del Governo, anche perché avete potuto svolgere il vostro intervento.

per quanto riguarda i lavori in Commissione, l'approvazione delle risoluzioni preclude il voto alle altre risoluzioni: questo vale per le risoluzioni come per i pareri alternativi. Quindi, non è vero e non può essere accolta l'interpretazione proposta dal senatore De Falco che sia stato in qualche modo precluso il voto sulla risoluzione in Commissione. La seconda questione è che per poter discutere le risoluzioni in Aula ci sono due condizioni: la prima è che sia approvata in Commissione, la seconda è che venga proposta da un terzo dei componenti la Commissione. Quindi, qualora non fosse proposta da un terzo dei senatori, non sarebbe sufficiente l'approvazione in Commissione, ma devono esservi entrambe le condizioni e da una lettura attenta dell'articolo 50 del Regolamento non sono assolutamente ammesse altre interpretazioni. Senatore De Falco, la pregherei, prima di far intervenire gli assistenti, di abbassare il cartello, anche perché sto rispondendo a lei. a lei. Chiedo agli assistenti di ritirare il cartello. Completo per dirle, senatore De Falco, come lei sa, che invece il testo della risoluzione è stato ammesso come ordine del giorno.

comprendiamo l'auspicio di colui che è seduto oggi ai banchi del Governo al posto del Presidente del Consiglio. Forse lo auguriamo a lui, ma non agli italiani

uno *stop* a ciò che sta accadendo, noi possiamo fare un'azione molto concreta e rapida. Dobbiamo sicuramente bloccare le partenze e dobbiamo fare in modo che il Mediterraneo non si trasformi in un obitorio a cielo aperto. Per fare questo, dobbiamo controllare i nostri confini.

Intanto, non riusciamo a seguire il suo intervento. Nonostante l'invito ai senatori ad abbandonare i banchi del Governo, questo non viene osservato. Inoltre, ci sono assembramenti sempre vicino ai banchi del Governo.

ore 17,30)*. Credo che possiamo riprendere i nostri lavori. Abbiamo dato esauriente conto della richiesta di spiegazioni sull'*iter* regolamentare:

o no. Avevamo interrotto il senatore Aimi, al quale chiediamo ovviamente scusa. Aveva parlato per pochi minuti; gli restituiamo la parola, restituendogli anche integralmente il tempo che aveva a disposizione. Prego, senatore Aimi.

siamo una grande potenza. La presenza dell'Italia nelle missioni internazionali come secondo contributore è la dimostrazione più palmare ed evidente dell'importanza che riveste l'Italia all'interno dello scacchiere internazionale.

reduci da discussioni estremamente delicate, che hanno dimostrato come l'Italia si riveli particolarmente fragile in questo momento. È un momento in cui soffiano venti di guerra, che soffiavano già un anno fa.

ci ha ammonito e ci ha chiesto se ci rendiamo conto di ciò che sta avvenendo nel giardino di casa nostra. Sta avvenendo ancora in queste ore in Iran, dove domani ci sarà

soprattutto in Algeria, ma non meno in Tunisia, dove c'è una situazione davvero drammatica e tante sono le partenze da quei lidi. In questo quadro, vedete, c'è anche tutta la dimostrazione della debolezza della politica europea. Un'Europa che non si è fatta superpotenza e un'Italia comunque forte, ma che non riesce a esprimere, se non con queste missioni, la sua vera e straordinaria natura. Siamo un popolo, comunque la si pensi, davvero straordinario e generoso; questo lo dobbiamo riconoscere. *(Applausi)*. La politica che vuole attuare Forza Italia è quella di mettere al centro, soprattutto in questa discussione,

in Africa e sei in Europa. Stiamo collaborando con le Nazioni Unite e con l'Alleanza atlantica, in un impegno davvero straordinario e lo dico a coloro che hanno i più alti incarichi di responsabilità. Per questo voglio ringraziare il Governo e in particolare il nostro sottosegretario

armate. Se vogliamo dunque provare a realizzare qualcosa di positivo, non possiamo dimenticare che il nostro orizzonte deve essere quello di una politica internazionale che guardi ai Paesi occidentali, come aveva indicato a Pratica di mare lo stesso presidente Berlusconi, quando aveva evidenziato che dobbiamo rimanere all'interno del perimetro dell'alleanza con l'occidente, che guardi

una data per noi straordinariamente importante, soprattutto perché segna un momento di riavvicinamento dell'Italia e degli italiani alla patria. In queste missioni internazionali abbiamo avuto più di 500 morti

i nostri paracadutisti della Brigata Folgore, di stanza ad Herat, sono rientrati, non abbiamo avuto uno spettacolo particolarmente edificante. È vero che c'era la pandemia, ma chiedo al Governo che si

la Marina militare, l'Aeronautica, ovvero l'Arma azzurra, i paracadutisti e l'Esercito. Pochi mesi fa ricorreva il 160° anniversario della fondazione

di Forza Italia alle nostre Forze armate e, dopo aver rivolto un pensiero commosso alla memoria di tanti, anch'io non posso non valutare ciò che sta avvenendo in queste ore in Afghanistan. Ci sono territori che vengono completamente devastati dall'arrivo dei talebani e abbiamo visto quest'oggi filmati terribili. Ci sono posti di blocco in cui le persone vengono esecutate sommariamente, magari perché indossano un abito all'occidentale. Abbiamo visto scene di decapitazione negli stadi: è un fiume di sangue che scorre, al quale dobbiamo porre fine e al quale dobbiamo davvero tutti insieme, in quest'Aula, dedicare grande attenzione. *(Applausi)*. Occorre uno sforzo importante da parte del Governo per fare sì che possa esserci il rientro di tutti coloro che hanno collaborato con le Forze armate italiane. naturalmente a tutti gli afghani che hanno avuto il ruolo di interprete, persone che si sono battute, molte delle quali sono state addirittura ferite in combattimento. Un'Italia grata ai propri militari non può essere ingrata nei confronti di coloro che hanno contribuito a salvare, per quello che era possibile fino a quel momento, la pace in quei territori. Non ci è piaciuto, naturalmente, il ritiro

Prima di arrivare alla mia conclusione, vorrei dire che questa Assemblea può fare tanto; soprattutto ha il dovere ha il dovere di ricordare i tanti che sono caduti. Vorrei solo, se me lo consente, Presidente, ricordare l'ultima medaglia d'oro:

nonostante fosse ferito, per andare a recuperare due ragazze, due commilitoni, che erano rimaste all'interno del blindato. *(Applausi)*. Questi sono i bellissimi esempi ai quali anche la migliore gioventù italiana dovrebbe rifarsi, non a quelli di chi pensa di erigere monumenti ai disertori o magari immagina un'Italia diversa. Abbiamo ancora bisogno di eroi, militari ma anche civili.

anche quest'anno, sempre con un po' di ritardo, ci apprestiamo a discutere in Aula l'autorizzazione per la partecipazione italiana alle missioni militari internazionali. Vorrei fare Vorrei fare due premesse prima di affrontare alcune questioni relative al tema in esame. La prima premessa che dobbiamo ricordarci, e questa è è una cosa che come Gruppo teniamo a rimarcare spesso, è che le Forze armate italiane sono uno dei fiori all'occhiello del nostro Paese. Va anche il mio ringraziamento al nostro sottosegretario, senatrice Pucciarelli, per il lavoro che sta svolgendo in questo momento. In un periodo di rinnovamento come questo in cui viviamo, cui si parla di riprogrammare il Paese da qui ai prossimi trent'anni, mettiamoci bene in testa che le nostre Forze armate devono essere considerate al pari delle altre eccellenze italiane. Le nostre Forze armate e in generale l'intero comparto della difesa italiano sono un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, un motivo di vanto per il nostro Paese e un *asset* strategico che ci permette di essere competitivi su scala globale. Arriviamo alla seconda premessa: le missioni internazionali non sono un grande carro al quale unirsi per motivi di opportunità politica, politica, ma rappresentano, soprattutto per una media potenza come la nostra, l'occasione che uno Stato ha per posizionarsi nel mondo; l'occasione, in sintesi, di perseguire i nostri interessi strategici internazionali, inseriti in un contesto multilaterale e di alleanze ben chiaro. Per tali ragioni è importante che il dibattito in Parlamento, la casa della democrazia *(Applausi)*, riscopra il valore altissimo perseguire gli interessi del nostro Paese, ma questo particolare viene troppo spesso dimenticato nei dibattiti politici che accompagnano la votazione delle missioni internazionali. Discorsi che derivano da una ideologia politica dovrebbero essere tenuti ben a distanza in tale sede di discussione: l'unico faro che dovrebbe accompagnare una votazione del genere è quello, come detto, del perseguimento dei nostri interessi nazionali, perché a questo serve lo strumento militare all'estero. Finite le premesse, vorrei analizzare velocemente alcuni aspetti estremamente positivi delle missioni internazionali che ci apprestiamo a votare. L'aspetto che mi preme sottolineare (e del quale sono pienamente soddisfatto) è quello che vede il quadrante africano, con ben 17 missioni, come prioritario per i nostri interessi. Continua la strategia che vede il nostro Paese aumentare la concentrazione delle proprie risorse verso il fronte Sud e verso quella parte del continente africano che si sviluppa all'interno del triangolo Golfo di Guinea, Corno d'Africa e Libia. Il continente africano è fondamentale per il futuro del nostro Paese, cari colleghi, prima di tutto nella regione nord-africana e saheliana, un'area prioritaria in termini di sicurezza e di contenimento dell'immigrazione clandestina. Siamo contenti che con l'avvento del nuovo Governo si sia finalmente tornati ad impegnarsi in maniera costante nella partita libica. Nord Africa e Sahel sono aree cruciali per il transito dei flussi migratori diretti verso il Mediterraneo e negli ultimi anni hanno vissuto un contesto di progressivo deterioramento della situazione di sicurezza e di profonda destabilizzazione dovuta a molteplici cause: dall'attivismo di gruppi armati jihadisti, ai conflitti interetnici e all'estrema povertà,

rapporti bilaterali con gli Stati. Una seconda regione africana fondamentale per gli interessi del nostro Paese è quella del Golfo di Guinea. caso i nostri interessi sono chiaramente di tipo energetico-commerciale: l'estrazione e l'approvvigionamento di idrocarburi, in relazione alla nostra industria, è il principale *asset* da tutelare. Bisogna ricordare che il 90 per cento circa dei sequestri in mare nel mondo sono avvenuti in quest'area, pertanto risulta fondamentale garantire la sicurezza delle rotte del commercio marittimo in questa regione e giungere a solidi rapporti bilaterali con Paesi come il Togo, il Benin, il Camerun, il Gabon, la Guinea equatoriale e il Congo, al fine di tutelare i nostri interessi commerciali a lungo termine. terza regione è quella del Corno d'Africa, che tra le altre cose presenta anche l'unica novità, insieme alla missione presso lo stretto di Hormuz, tra le missioni per il 2021. Parlo chiaramente della nuova missione in Somalia, dove un rappresentante italiano prenderà parte alla United Nations assistance mission. Siamo contenti che il nostro Paese, insieme alle organizzazioni internazionali, dimostri di voler continuare a lavorare per il rafforzamento delle Istituzioni somale e del Governo federale di transizione. Il Corno d'Africa, un tempo quadrante nel quale la nostra capacità di proiezione e influenza era prima nel mondo, rimane un'area prioritaria per gli snodi commerciali globali e l'Italia ha il dovere di giocare un ruolo di primo piano. Per concludere, mi sia consentita una rapida menzione all'annuncio della guida italiana della missione in Iraq. un importante riconoscimento per un impegno ventennale, che va onorato anche nel ricordo dei militari italiani che hanno perso la vita combattendo il terrorismo e cercando di stabilizzare un Paese dilaniato da guerre e povertà. *(Applausi)*. Ci siamo impegnati in Afghanistan, dimostrando grandi capacità dal punto di vista addestrativo e della vicinanza alla popolazione, e faremo sicuramente Abbiamo un capitale da spendere, grandi capacità e una grande credibilità maturata nei confronti degli alleati. L'Iraq è un Paese da ricostruire e assumere la *leadership* della missione militare vuol dire favorire il nostro coinvolgimento nella fase di ricostruzione. Questo è quello che intendiamo con l'utilizzo dello strumento militare come capacità di posizionarsi nel mondo: sinergia tra il mondo della difesa, quello quello economico e quello diplomatico. Questo è quello che serve al nostro Paese per riaffermarsi nel prossimo futuro come uno dei principali attori dell'Alleanza atlantica.

anche per noi del MoVimento 5 Stelle il ritardo con cui la deliberazione è stata presentata alle Camere va stigmatizzato, in quanto limita l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e indirizzo politico su una materia cruciale come la politica militare internazionale. E questo è tanto più grave quando si parla di missioni che vengono sospese, o mutano radicalmente la loro natura nel corso dell'anno prima del passaggio ai due rami del Parlamento.

Fatta questa premessa, entriamo nel merito della questione mettendo subito in chiaro che per il MoVimento 5 Stelle la tutela dei diritti umani rimane un obiettivo irrinunciabile e imprescindibile sempre e ovunque e anche in Libia, dove i nostri obiettivi primari consistono nell'assicurare la sicurezza e il processo verso la stabilità nazionale. Faremo ciò condividendo le nostre competenze in ambito sanitario, rafforzando la sicurezza, fornendo assistenza specialistica nell'addestramento delle milizie, monitorando e anticipando con l'azione diplomatica le criticità che possono dar vita a nuovi episodi di *escalation* militari in cui - ricordiamolo - è sempre la popolazione locale a pagare il prezzo. A differenza di quanto riportato in un intervento di chi mi ha preceduto, ci tengo a precisare a gran voce che il Governo italiano non ha disposto finanziamenti a favore della guardia costiera libica. *(Applausi)*. Lo dico per evitare che si diffondano notizie false e tendenziose. È chiaro che c'è ancora tanto da fare ed è doveroso da parte dell'Italia esserci. In proposito, ricordo che qualche settimana fa, per la prima volta nella storia, proprio qui in Italia abbiamo accolto la coalizione anti-Daesh, un evento che testimonia concretamente quanto si stia facendo per contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale; evento che testimonia il grande impegno del ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, al quale poi sono state indirizzate delle pesanti minacce pubblicate dal settimanale dell'ISIS «Al-Naba». Ma il processo di stabilizzazione dell'area deve continuare. L'Italia deve essere il perno centrale del Mediterraneo fino a che tutte le operazioni non saranno condotte sotto la guida dell'Unione europea, fino a che l'Europa non si farà carico della formazione e del supporto alla Guardia costiera libica. Fino a quel momento, l'Italia non può tirarsi indietro. Infatti, se decidessimo di staccare la spina, si creerebbe un corto circuito pericoloso, un incremento esponenziale dei flussi migratori con barconi e carrette del mare con a bordo uomini, donne e bambini, che partirebbero dalle coste per navigare in condizioni disumane mettendo a repentaglio la propria vita. Questo non deve più accadere. Tutte le iniziative messe in campo volgono proprio in questa direzione, quella della tutela delle condizioni degli esseri umani, di favorire una gestione più efficace degli standard internazionali dei flussi migratori, garantire protezione ai più vulnerabili e contrastare quindi il traffico degli esseri umani. Non meno importante però è far notare che il vuoto determinato dalla nostra assenza permetterebbe ad altri Paesi - che non aspettano altro - di intrufolarsi, producendo grave pregiudizio per il ruolo futuro che il nostro Paese potrà svolgere in Libia. In tema di cooperazione per il controllo dei flussi migratori e di Nord Africa, non posso non esprimere forte preoccupazione per la situazione in Tunisia, Paese di primaria importanza da questo punto di vista, sul quale l'Italia sta conseguentemente investendo molto. La crisi politica tunisina rischia di aggravare ulteriormente una situazione socioeconomica già critica, che sta spingendo un'intera generazione di giovani tunisini a lasciare il Paese. Per non parlare delle pericolose ripercussioni della crisi politico-istituzionale sulla funzionalità e l'operatività delle autorità tunisine preposte al controllo delle acque costiere. Il rischio è un incontrollato *boom* di partenze di barconi. È urgente ripristinare la stabilità politica, economica e sociale della Tunisia, anche implementando tutti gli interventi della cooperazione italiana previsti dall'ultimo *memorandum* d'intesa sulla cooperazione italo-tunisina a sostegno dell'occupazione giovanile, dell'istruzione e dello sviluppo. Rimanendo in tema di cooperazione con l'Africa, anche in chiave di contrasto alle cause dei flussi migratori, l'altra situazione che desta forte preoccupazione è quella dell'Etiopia, dove la crisi umanitaria scatenata del conflitto del Tigray assume una dimensione drammatica con centinaia di milioni di persone sfollate all'interno dello stesso Paese e delle vicine regioni di Afar e Amara, mentre oltre 60.000 rifugiati hanno già attraversato il confine con il Sudan. È urgente che l'Etiopia garantisca l'accesso umanitario a queste regioni per scongiurare il peggio. Considerando che il nuovo programma triennale di cooperazione italiana con l'Etiopia è ancora in fase di definizione, riteniamo doveroso modulare tutti gli interventi di cooperazione verso questo Paese alla luce di quanto sta accadendo. Veniamo al Paese che più a lungo ha impegnato le nostre Forze armate

Un costo umano ed economico altissimo per una missione di cui il MoVimento 5 Stelle ha sempre chiesto la conclusione con il ritiro dei nostri soldati: rammento a tutti che questa è stata la prima richiesta politica presentata con una mozione che il MoVimento 5 Stelle ha fatto appena entrato in Parlamento nel 2013. Oggi quindi non possiamo che essere felici per la conclusione di questa ventennale spedizione militare, ma non possiamo essere altrettanto soddisfatti per il modo in cui si sta concludendo. Pur di non riconoscere la fallimentare realtà di questa guerra, con i talebani rimasti al potere in quasi tutto il Paese e un Governo instabile, che senza le truppe NATO, non controlla nemmeno Kabul, si è deciso di abbandonare il campo nella pia illusione che lo sgangherato esercito afgano riesca a resistere da solo. Non si è voluto, prima di levare le tende, trattare veramente con i talebani, che rappresentano la maggioranza pashtun della popolazione, per includerli in un nuovo futuro governo federale e multietnico, a patto del loro impegno contro ISIS e al-Qaeda e per il rispetto dei diritti umani e delle donne. Una soluzione che, per inciso, i talebani si dicono ancora oggi pronti ad accettare in cambio del cessate il fuoco. Per non vanificare gli sforzi fatti e i risultati ottenuti e per non lasciare sprofondare l'Afghanistan in una nuova guerra civile, come MoVimento 5 Stelle auspichiamo che l'Italia si faccia promotrice di una vera missione di *peacekeeping*, rimanendo in prima linea con una missione civile, che lavori intensamente per la riconciliazione nazionale e il disarmo delle milizie, per la ricostruzione del Paese e per rafforzare la cooperazione allo sviluppo, per la tutela dei diritti umani. Concludendo il mio intervento, signor Presidente, mi permetto di fare una considerazione e un ringraziamento. La considerazione, positiva, riguarda l'incremento degli stanziamenti finanziari per garantire sicurezza e protezione ai nostri diplomatici e connazionali in Paesi a rischio, un'esigenza fondamentale, che purtroppo viene spesso dimenticata per tornare alla ribalta solo a seguito di fatti drammatici, come l'assassinio avvenuto in Congo lo scorso febbraio del nostro giovane ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista locale. Un ringraziamento va ai nostri Ministri, al ministro della difesa Lorenzo Guerini e al ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, impegnati nella costante attività e trattazione dei rapporti internazionali per proseguire il dialogo per il processo di stabilizzazione e favorire al meglio lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre prossimo, l'attuazione del cessate il fuoco, l'adozione del bilancio unificato, la riconciliazione nazionale. Infine, dal momento che l'Italia partecipa a ben 40 missioni internazionali, voglio rivolgere al personale civile e militare e alle loro famiglie, alle componenti delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, a tutti gli uomini e le donne impegnati per l'Italia in tutti i teatri operativi. A loro va il ringraziamento per tutto ciò che fanno e per come lo fanno. Grazie a voi, che rendete l'Italia grande nel mondo.

grazie a tutte

ho presentato è perfettamente compatibile e coerente con i contenuti del decreto; non c'è nessun problema di inammissibilità buon intenditore, poche parole. Chiedo quindi alla Presidenza la possibilità di riaprire i termini per depositare un ordine del giorno che volentieri condividerò con i colleghi che intendano sottoscriverlo.

La ringrazio molto,

attenta, appassionata e anche critica, tenevo a replicare brevemente su uno dei punti che sono stati più volte richiamati, che è quello che riguarda l'Afghanistan. Come sapete, il ritiro è stato deciso secondo il principio *in together, out together* e non vogliamo che segni la fine del sostegno internazionale al Paese, soprattutto alla luce del rapido deterioramento deterioramento della situazione sul terreno, e continueremo a sostenere la popolazione e le istituzioni afghane con un rafforzamento della cooperazione civile. Rispetto a un tema che avete sollevato, onorevoli senatori, il Ministero della difesa e la Farnesina stanno lavorando per trasferire quanti in questi anni hanno collaborato con il nostro contingente e con i loro familiari. Con l'Operazione Aquila si sta organizzando il trasferimento umanitario del personale civile afghano che è stato al fianco dell'Italia. Ad oggi sono giunti in Italia 228 tra collaboratori e loro familiari; hanno già concluso la quarantena e sono stati ricollocati sul territorio nazionale. Tra agosto e ottobre la Difesa conta di completare un secondo rientro che dovrebbe riguardare circa 400 cittadini afghani la Farnesina sta lavorando a misure per facilitare il trasferimento in Italia dei cittadini afghani che hanno collaborato con l'ambasciata e gli uffici della cooperazione allo sviluppo. È un impegno morale e fattivo, che vede coinvolti i Ministeri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, come segnale che non intendiamo abbandonare chi ha lavorato per la libertà e la democrazia in Afghanistan. che stiamo considerando - insieme agli altri *partner* dell'Unione europea - iniziative sotto l'ombrello delle Nazioni Unite sia a New York che a Ginevra che prevedano meccanismi internazionali volti a monitorare per prevenire massicce violazioni dei diritti umani. Si tratta di iniziative naturalmente da prendere

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto

Forza Italia ritiene che le missioni militari internazionali siano un'occasione per qualificare l'impegno dell'Italia in favore della democrazia, del diritto dei popoli, della pace e della libertà. Riteniamo che le missioni militari di pace siano anche uno strumento di politica internazionale e che, non solo nell'area mediterranea, ma anche negli altri luoghi, ben più lontani, dove siamo tradizionalmente presenti, siano sempre state motivo di orgoglio, di onore

però, il dibattito c'è, com'è normale che sia, perché il Regolamento consente di attivare questa procedura, cogliamo l'occasione non solo per ribadire tale posizione, grazie a tutte alla capacità con cui stanno operando in contesti spesso ancora attraversati da conflitti e da fenomeni di terrorismo, dimostrando la capacità italiana di educare alla democrazia, al dovere e alla gestione corretta dei territori e del governo dei popoli. Tuttavia, il ritardo con cui si discute di queste materie ci pone di fronte a un dilemma. Stiamo per votare la prosecuzione della parte finale della missione in Afghanistan, che in realtà si è conclusa, perché poi i provvedimenti arrivano un po' sfasati;

In quest'Aula è stato sollevato il tema degli interpreti, persone che hanno collaborato con gli italiani, con gli americani e con le truppe della NATO e che oggi sono esposte alla ritorsione dei talebani. Non è solo questo il problema, però, cari colleghi: si tratta un dovere morale, perché in un Paese in cui sbarcano clandestinamente persone che non hanno alcun diritto di venire qui credo che sia doveroso accogliere chi si è sacrificato insieme a noi per la libertà del proprio popolo. abbiamo posizioni chiare, ma non ci si può limitare al tema degli interpreti. Leggete le cronache: ho qui articoli che fino a questa mattina ci raccontano di come oramai il dominio talebano in Afghanistan sia arrivato all'85 per cento del territorio; i talebani cominciano a riconquistare le città,

In un momento in cui ci sono fenomeni gravi di migrazione, avremo una situazione molto drammatica, che si potrebbe abbattere sull'Occidente. I talebani, com'è stato già detto, hanno contatti con la Cina e ci sono pericoli anche sotto il profilo geopolitico. Qui facciamo un gran parlare di diritti, abbiamo sospeso la discussione di una controversa legge, ma i diritti delle donne afghane e di coloro che subiscono la dittatura talebana, li vogliamo ricordare o li dobbiamo archiviare? archiviare? A quelli che vorrebbero farci approvare leggi un po' discutibili su altri campi ricordo che i diritti vanno osservati a 360 gradi. Abbiamo partecipato alla missione afghana dopo l'11 settembre, perché l'Afghanistan era il luogo da cui più partivano le offensive contro il mondo e dove, da Bin Laden ad altri, hanno trovato rifugio - in complicate zone montuose, che né gli inglesi, né i russi, né altri nel corso dei secoli sono mai riusciti a controllare, quelli che un tempo chiamavamo i *mujahidin*, quando si opponevano all'invasione russa, e che poi, presi dal fondamentalismo, si sono rivelati una minaccia per il mondo libero. Penso che dovremmo riflettere se sia stato opportuno interrompere quella missione. Del resto, il disimpegno americano - diciamoci la verità - non consentiva ad altri Paesi di rimanere lì, perché la forza e l'organizzazione degli Stati Uniti è comunque uno scudo anche per le missioni multilaterali e internazionali e quella afghana non è stata una passeggiata. Stanno forse per espugnare Herat: ve lo ricordate questo nome, Herat? Vi era una posizione degli italiani. Abbiamo sacrificato fatica e sangue per difendere quella terra, che oggi sarà espugnata. È solo un problema di tempo. Poi leggo che l'attuale Governo afghano manda truppe e non so cosa intenda fare, ma credo che non ci sia confronto. ci sia confronto. Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo, ma mi rendo conto di non poter sovraccaricare i Sottosegretari qui presenti di un problema planetario: penso che forse la comunità internazionale si dovrebbe interrogare. Non sono qui a chiedere voti per parti separate, perché condividiamo l'impegno in Libia e riteniamo che chi intende disarmarlo voglia favorire ulteriore immigrazione clandestina in Italia. *(Applausi)*. Preoccupiamoci degli interpreti afgani, non dei clandestini che dalla Libia vengono in Italia.

I temi del fondamentalismo non sono infatti esauriti: riaffiorano, ora qui, ora là, e anche la crisi della Tunisia, un Paese che sta a poche miglia dalla Sicilia, contiene questo germe. È inutile che facciamo finta di non accorgercene. I fenomeni del Nord Africa, la presenza turca e tanti altri fattori ci fanno capire che forse, cari colleghi, non solo dobbiamo confermare queste missioni e ovviamente anche la scheda n. 48, ma semmai augurarci che l'Italia possa istruire sempre di più la Guardia costiera libica sostenere la Libia verso un cammino di democrazia e di libertà, come fecero i governi Berlusconi (e oggi si sono dovuti recuperare i Patti di amicizia tra l'Italia e la Libia). Ricordo quelli che ridevano per le tende a Villa Pamphili: si preoccupassero degli accampamenti di clandestini che ci sono in tutta Italia. Dialogare con Gheddafi forse dava più frutti che inseguire situazioni di instabilità. instabilità. Pertanto, nel confermare tutte le missioni e nel rinnovare la solidarietà e il sostegno alle Forze armate, voglio anche ringraziare il ministro Brunetta.

dignità alle missioni internazionali, che tanta parte sono della politica estera e dell'immagine dell'Italia nel mondo, proprio venendo a discutere di questo documento così importante e di questa risoluzione in Parlamento.

Chi presiede quest'Assemblea è stato Ministro della difesa e sa, come e meglio di noi, che la pietra angolare della politica dell'Italia nel mondo sono le missioni internazionali. insieme ai nostri militari, donne e uomini, con un aiuto collaterale e parallelo del volontariato di forze straordinarie che l'Italia mette in campo, sono sono l'immagine emblematica di quello che gli italiani fanno per gli altri, in modo originale, con competenza e con professionalità.

e la situazione rischia, purtroppo, di riportare le lancette dell'orologio a vent'anni fa. Quello che sta capitando - al di là dei colloqui di Doha degli approcci con l'amministrazione americana di Trump e poi di Biden - tra i talebani e gli occidentali è stato, in gran parte, un cumulo di parole e di impegni scritti sulla sabbia.

che la comunità occidentale, a partire dall'Europa, dall'Italia e dagli Stati Uniti, si deve interrogare su quello che è stato, oggettivamente,

abbiamo consentito l'accesso all'istruzione delle ragazze afghane, che erano obbligate a fare le serve in casa. Tutto questo è un risultato che non può essere macchiato da un ritorno *sic et simpliciter* a vent'anni fa. Il rischio c'è, Il rischio c'è, perché un'interpretazione fuorviante e tradizionalista dell'Islam, come alcuni fanno in quella realtà, rischia di azzerare la battaglia per i diritti civili che è stata fatta. Non è stata fatta una battaglia contro i talebani, per un problema solo di contrasto al terrorismo. Vi ricordate quando i talebani buttavano giù monumenti che erano patrimoni di culture che

anche in Afghanistan in condizione di avere diritto di cittadinanza. Bene, colleghi, il discorso è troppo complicato e non posso continuarlo, perché siete tutti troppo intelligenti e avete capito quello che voglio dire. Prima di trovarci un nuovo Afghanistan negli anni prossimi, mi auguro che la comunità occidentale rifletta bene, perché rischiamo di avere, dall'Afghanistan all'Iraq, lo stesso scenario che drammaticamente si ripete. Libia, sono un grandissimo estimatore del collega Verducci, che peraltro collabora con me, come vice presidente, nell'Unione interparlamentare. Non condivido evidentemente il suo ordine del giorno, ma voglio anche dire che comprendo quello che egli esprime. D'altronde, una una garanzia dal punto di vista della nostra politica estera, come Emma Bonino, ha avuto molte considerazioni analoghe a quelle che fate. Colleghi, il punto però, anche qui, come sull'Afghanistan, è che dobbiamo guardarci in faccia e dire con realtà che stiamo trasferendo sul mare un problema di terra.

Perché siamo inefficaci sulla terra e perché abbiamo perso qualsiasi possibilità di incidere sul tema libico, come rischiamo di averla persa sul tema della della Tunisia, perché è in corso nel Mediterraneo una guerra non dichiarata, ma combattuta aspramente tra il Qatar e la Turchia, da un lato,

che affermiamo votando queste missioni internazionali di pace. Qui allora c'è da ripensare tutto e da ripensarlo fuori dagli *slogan*. Abbiamo avuto la retorica pro-Trump e quella anti-Trump; la realtà delle cose è che la politica di Trump oggi - a parte le buone maniere e una capacità di una capacità di stare al mondo leggermente migliore - non credo sia molto smentita da quello che sta facendo Biden, ad esempio negli approcci sul multilateralismo e sull'Europa. Questo è un problema per noi, perché dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. L'Italia è l'unico Paese e l'unico azionista del Mediterraneo che è riuscito, allo stesso momento, a essere contro l'Egitto e contro la Turchia, che sono grandi nemici tra di loro nel Mediterraneo. Scusate, ma allora qualche problema ci sarà nella nostra politica. Probabilmente

di non pagare questi *sentiment* e che non ci sia qualcuno che sta giocando sul sentimento nazionale che l'Italia giustamente rivendica per sostituirsi a lei sotto altri profili. Qui c'è un groviglio e il tema delle missioni internazionali di pace è la goccia rispetto a un tassello e a un mosaico che non riusciamo più a governare. Colleghi, votiamo queste missioni, ma credo che abbiamo veramente tanto da fare, per cercare di capire lo scenario geopolitico in cui ci muoviamo, ci muoviamo, pieno di preoccupazioni e che, a mio parere, consegna a voi e ai nostri figli un Paese e una situazione internazionale molto più difficili.

di aver risolto la metà dei nostri problemi. Il risultato è che i problemi si sono aggravati e oggi ce ne troviamo ancora di più. Credo che, in termini geopolitici, abbiano molte riflessioni da fare soprattutto coloro che hanno la responsabilità di gestire il Governo del Paese.

pace e stabilità sul fronte internazionale e sicurezza per le donne e gli uomini dei nostri contingenti, oltre che sul fronte interno: questi sono gli obiettivi con i quali ci apprestiamo oggi a votare il rinnovo delle nostre missioni internazionali. Esse si sviluppano su un doppio binario: il nostro impegno al fianco della NATO, nel solco di un'Alleanza atlantica finalmente rinsaldata senza ambiguità, grazie al nuovo Esecutivo, e dall'altro lato le missioni europee, necessarie per favorire processi di normalizzazione geopolitica, in una serie di territori strategici anche per la nostra sicurezza interna. Nel complesso, a parte il ritiro dall'Afghanistan, per l'anno in corso il decreto missioni va sostanzialmente a confermare le missioni internazionali già in atto nel 2020 in tre continenti, con una progressiva attenzione al Mediterraneo allargato, perseguita anche con l'avvio di due nuove operazioni: una prima nello Stretto di Hormuz, con l'impiego di un dispositivo aeronavale rivolto soprattutto al contrasto della pirateria a danno di navi commerciali, ed una seconda operazione in Somalia, con un nostro dispiegamento volto a favorire la promozione dello Stato di diritto. I nostri impegni operativi nell'area africana si evolvono quindi con numerose missioni italiane, a conferma di una strategia che si pone l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione nei confronti del Continente africano, in particolare nell'area compresa nel triangolo tra il Golfo di Guinea, il Corno d'Africa e la Libia al Nord. Soprattutto in Libia riteniamo che sia necessario restare e che il nostro Paese debba essere protagonista attivo nel processo di stabilizzazione, attraverso un impegno che miri anche ad arginare l'irruente protagonismo di forze straniere esterne, che cercano di approfittare della fragilità libica, per dare voce alle proprie mire espansionistiche. Un nostro allontanamento vorrebbe dire creare ulteriore instabilità nel Mediterraneo. Noi invece ribadiamo la necessità che la nostra presenza in Libia debba servire alla tutela dei diritti umani, perché non è tollerabile che la guardia costiera locale speroni gommoni con migranti a bordo o spari ai pescherecci dei nostri pescatori ed è ancora meno accettabile che lo faccia se viene finanziata e formata dal nostro Paese. Non possiamo sopportare che violazioni del diritto internazionale di questo tipo possano avvenire con l'avallo dei nostri soldi pubblici. Già lo scorso anno, in occasione del voto sulle missioni internazionali, il Governo italiano si era impegnato ad intervenire nei confronti della Guardia costiera libica, allo scopo di indurla al rispetto dei diritti umani ed internazionali. Il Governo aveva infatti accolto un nostro ordine del giorno, sottoscritto da diverse forze politiche, che prevedeva corsi di formazione ai libici tarati sul rispetto dei diritti umani, il libero accesso di organizzazioni internazionali ai centri di accoglienza e la previsione di corridoi umanitari per un'immigrazione legale. Ad un anno di distanza, però, questo impegno resta purtroppo in gran parte disatteso e la situazione è ulteriormente peggiorata, come dimostra la cronaca delle ultime settimane. È per questo che la settimana scorsa in Commissione affari esteri, emigrazione e oggi qui in Assemblea chiediamo la votazione del provvedimento per parti separate, rispetto alla scheda inerente i finanziamenti alla Guardia costiera libica, finanziamenti sui quali, come Italia viva, non prenderemo parte al voto. Il nostro intento è infatti quello di esprimere due considerazioni politiche. esprimiamo la nostra ferma volontà di sostenere convintamente le missioni internazionali, che riteniamo debbano essere un chiaro momento di unità nazionale al fianco delle nostre Forze armate. Al tempo stesso, però, sentiamo l'esigenza di segnalare il nostro disappunto rispetto alla missione in questione. Se da un lato siamo contrari al disimpegno dell'Italia dalla Libia, dall'altro lato siamo convinti che la nostra presenza debba servire alla salvaguardia dei diritti e non a violarli. Riteniamo quindi che sia doveroso interrogarsi su come rimodulare il nostro impegno a sostegno della Guardia costiera libica, onde evitare che i nostri finanziamenti finiscano nelle mani sbagliate a favore di torturatori ed aguzzini. aguzzini. Proprio perché crediamo fortemente nel ruolo dei nostri contingenti, non parteciperemo al voto sulla scheda n. 48. Con il provvedimento al nostro ordine del giorno l'azione italiana si esercita anche nel quadrante mediorientale asiatico nella regione del Golfo persico, dove il nostro Paese è presente con diverse missioni, a partire dal Libano, un territorio in cui permangono un preoccupante stallo istituzionale ed una costante decrescita economica, che rischiano di portare il Paese al collasso. Ecco perché l'Italia conferma il suo impegno accanto alle forze di sicurezza libanesi ad un anno esatto, oggi, dalla terribile esplosione al porto di Beirut. Altrettanto strategica, in una chiave di lotta al terrorismo, ma anche di compartecipazione alla ricostruzione economica del Paese, è la conferma del nostro impegno italiano in Iraq, un Paese che da anni è tra i nostri primi fornitori di greggio. Ma con il rinnovo delle missioni internazionali perseguiamo l'obiettivo della lotta all'ISIS anche in altre aree, in particolare nel Nord Africa, nel Sahel, come pure nell'Africa subsahariana ed in Mozambico, dove la sicurezza è minacciata da affiliati di Daesh che sono stati capaci di ricompattarsi e rappresentano una concreta minaccia politica e militare e dove la nostra presenza su determinati territori può essere decisiva per ostacolare sul nascere tutta una serie di possibili cellule terroristiche. Viene inoltre confermata la nostra importante presenza in Niger, dove siamo dal 2018 con una missione bilaterale di supporto volta a contrastare il traffico di esseri umani verso la Libia, a conferma di quanto il nostro Paese si è impegnato sul fronte del contrasto alla criminalità internazionale ed ai fondamentalismi. Con il medesimo impegno è necessario che l'Italia operi per la pacificazione dell'Afghanistan, nonostante si sia appena conclusa la nostra missione ventennale, perché lasciare solo il popolo afghano vorrebbe dire pagarne presto probabilmente noi stessi le conseguenze. Per quanto riguarda invece il quadrante europeo, le nostre Forze armate sono presenti in sei missioni. In particolare resta cruciale quella nell'area dei Balcani, che purtroppo continua ad essere la polveriera storica d'Europa, dove l'eventuale acuirsi delle tensioni potrebbe avere effetti devastanti in tutta l'area e dove quindi è interesse diffuso garantire una maggiore stabilizzazione. Il rifinanziamento delle nostre missioni internazionali risponde anche alla necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza per i nostri militari. Sono 9.449 le donne e gli uomini impegnati nelle diverse operazioni in giro per il mondo, veri costruttori di pace che svolgono un ruolo prezioso anche per i Paesi nei quali operano, spesso provvedendo alla costruzione di strade, scuole, ospedali, attraverso un lavoro svolto con dedizione e senso dello Stato, in quegli stessi luoghi in cui fino a poco tempo prima c'erano solo bombardamenti e macerie. Si espongono però a rischi sempre più insidiosi, legati anche a nuove tipologie di minacce, le cosiddette guerre ibride, caratterizzate da molteplici tipologie di attacchi che richiedono adeguati livelli di difesa sia rispetto all'equipaggiamento che in termini di formazione e specializzazione. Ecco che si rende necessario raggiungere *standard* di capacità militari sempre più elevati, che consentano al tempo stesso di allinearsi a livello internazionale in un'ottica di una completa autonomia europea nel settore della difesa. Il dibattito sul decreto missioni può diventare quindi anche un'occasione per capire quanto ci sia bisogno di uno sviluppo delle Forze armate nazionali il più possibile coordinato ed integrato a livello europeo. Alle nostre porte abbiamo degli scenari geopolitici complessi, che mettono in pericolo la nostra sicurezza. Ecco perché serve una strategia comune di sicurezza nazionale ed estera che dia all'Italia e all'Europa la capacità di affrontare al meglio quelle situazioni conflittuali che abbiamo nella sfera geopolitica di nostro interesse. Conflitti che possono avere ripercussioni strategiche sul nostro Paese e sull'intero Continente in tema di approvvigionamento energetico, ma anche per la tutela da attentati terroristici o rispetto a flussi migratori. È necessario, quindi, che l'Italia si prodighi affinché l'Unione europea acquisti maggiore peso e protagonismo nella politica di difesa e di sicurezza e che diventi propulsore di politica estera a tutela degli interessi dell'intero Continente, non per diventare artefice di aggressioni, ma per essere in grado di essere attore di pace e non passivo spettatore delle guerre altrui. Tuttavia, il provvedimento sulle missioni internazionali è anche lo strumento più importante col quale il nostro Paese si confronta e contribuisce a questa complessiva strategia di difesa e sicurezza a livello internazionale, inoltre è l'occasione per il nostro Parlamento per ringraziare di cuore e per esprimere calorosa vicinanza

Fratelli d'Italia ha sempre votato a favore delle missioni internazionali e sarà sempre al fianco delle nostre Forze armate impegnate sia in Patria che all'estero. Pertanto neanche questa volta faremo mancare il nostro voto favorevole, ma diciamo con convinzione basta ai ritardi con cui

provvedimenti che si sono conclusi, missioni che si sono svolte, che sono finite. Insomma, la nostra è un'approvazione *ex post,* alla quale diciamo basta. È da tempo che Fratelli d'Italia richiede che su questa materia ci siano tempi puntuali e adeguati a confrontarsi sulle scelte di politica estera, fare un punto politico sulle missioni effettuate e anche sugli scenari più critici e anche così mutevoli. Tornando alla schizofrenia nella quale tutto questo accade, desidero anch'io citare la questione dell'Afghanistan. Noi oggi approviamo una missione che si è conclusa con il ritiro del nostro contingente

tra i primi ha denunciato con le sue interrogazioni, ovvero il rientro degli interpreti, delle loro famiglie, di coloro che hanno collaborato. Lei ha parlato di 228 rientri. Sono contenta perché a noi ne risultavano 182; è meglio così;

con gli Emirati Arabi Uniti. Si fa finta di niente e si continua a nascondere la testa sotto la sabbia. Abbiamo anche interrogato i Ministri competenti perché ci risulta - ed è noto - che siamo stati sloggiati dalla nostra base aerea di Al Minhad. Senza tanti complimenti, ci hanno mandato via e il 2 luglio abbiamo dovuto sbaraccare in fretta e furia. Naturalmente ci sono dei retroscena

Non abbiamo delle risposte neanche sul comando Irini, che ha atteso i visti per entrare a Tripoli. Probabilmente in Libia non ci vogliono e si preferiscono altre pressioni straniere extra-europee (penso alla Russia e, con preoccupazione maggiore, alla Turchia).

potrebbe essere una forza di controllo su tutta la rotta centrale del Mediterraneo, anche per prevenire il traffico di esseri umani ad opera degli scafisti. Ci sono tanti nodi che passano attraverso le autorizzazioni che diamo *ex post* - lo ripeto - alle nostre missioni internazionali. C'è anche la questione controversa della scheda n. 48, relativa all'addestramento della guardia costiera libica. Cerchiamo di

che per la condotta e la politica estera di questo Governo e di quelli che si sono succeduti in questa legislatura. Saremo sempre a favore delle nostre Forze armate perché

e italiana e la facciamo conoscere e apprezzare al resto del mondo. Nessuno ha mai potuto parlare male dei nostri contingenti e mai nessuno dei nostri militari si è macchiato di alcunché,

Quello che facciamo in missione tiene lontano dalle nostre case la minaccia terroristica e oggi più che mai questo è fondamentale. Parlavamo ieri di sfide della *cybersecurity*. Con le nostre missioni, missioni, come dicevo, portiamo una vocazione mediterranea, una identità precisa e una volontà di essere costruttori di pace. pace. Vorrei che la politica estera del Governo avesse una postura credibile, coerente, lineare, in grado di onorare gli impegni presi. Vorrei semplicemente che la politica estera del Governo fosse all'altezza

dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per i documenti così come presentati dai relatori. Stiamo parlando delle missioni internazionali, cioè della tutela del nostro interesse nazionale primariamente, cosa che sta a cuore alla Lega da sempre, e siamo con gratitudine al fianco delle nostre Forze armate. Dico questo perché nel dibattito è emersa una tendenza a parlare di ciascuna missione come fosse un qualcosa a sé. C'è, a mio avviso, un eccesso di analisi ma ci vuole invece una certa capacità di sintesi. Mi spiego meglio. Partendo da Ovest, troviamo missioni nel Golfo di Guinea (innanzi alle coste della Nigeria e della Guinea Equatoriale), missioni nell'Africa subsahariana; le missioni e gli interventi in Libia, nel Mediterraneo centrale, nei Balcani, nel Mediterraneo Orientale, in Libano, in Iraq e Siria, nella Penisola arabica, nel Golfo di Aden, nel Corno d'Africa, e lo Stretto di Hormuz è la novità di quest'anno. Ma che cosa vuol dire? dire? Se uniamo tutti questi puntini e guardiamo non alla singola missione ma al percorso, vediamo il percorso della nostra linfa vitale: l'energia. Siccome si parla sempre di fabbisogno di petrolio, di fonti energetiche e di materie prime, non si parla mai di numeri. Nel dicembre 2020 l'Italia ha avuto un fabbisogno, guardando solo al petrolio (escluso quindi il gas naturale), di 1 milione di barili al giorno. Un milione di barili sono circa 159 milioni di litri; ripeto, al giorno. Dallo Stretto di Hormuz, per fare una proporzione, passano 18 milioni di barili al giorno; dal Canale di Suez circa 1,5 milioni. Non Non stiamo parlando di ricchezza, ma di far funzionare il Paese. È per questo che invito a un maggiore pragmatismo nell'esame delle missioni internazionali, perché si rischia di confondere l'ideale con il reale

tra bersaglieri e carabinieri sbarcarono in Libano, sotto la guida dell'allora colonnello Tosetti. Ha un significato particolare, perché è stata la prima missione internazionale dopo la Seconda guerra mondiale. della difesa era Lelio Lagorio del Partito socialista, che si impegnò particolarmente per questa missione. certamente tutti parlano bene delle nostre Forze armate, del rapporto con le popolazioni locali, dell'apporto a livello di tutela dei diritti umani e difesa della democrazia, ma non dobbiamo dimenticare non è un gioco a punti; non stiamo dimostrando a qualcuno quanto siamo bravi. Dobbiamo tutelare i nostri interessi, il che non vuol dire fare un gioco da gioco da mercanti. Il problema è la sopravvivenza e il funzionamento del Paese. Visto che si parla di transizione ecologica,

il rapporto transatlantico è perno della nostra politica estera. Rifiuto infatti di pensare che ci sia qui dentro qualcuno eletto democraticamente che ritenga che la Cina sia il riferimento per la società del futuro

e oggi di nuovo a Biden, Presidenti che possono piacere o non piacere, a seconda dei gusti politici di chi siede qui, ma c'è stata l'alternanza. Xi Jinping non ha alternative, a meno che chiaramente non venga rinchiuso dal resto del partito in qualche campo di rieducazione per essere sostituito con un altro oligarca o autocrate che sia. Di conseguenza, è chiaro il nostro schieramento. Voglio sottolineare un altro aspetto. Si parla di multilateralismo e anch'io sono multilateralista, anche se gli "ismi" non mi piacciono. Sono un multilateralista molto moderato. Per me la NATO è il punto di riferimento e, quando si parla e si insiste a parlare di Unione europea in rapporto ai problemi dell'immigrazione nel Mediterraneo, mi sembra un po' come la mosca contro il vetro: non so se avete presenti quelle mosche che girano, che vogliono uscire, ma non vedono il vetro e continuano a sbatterci sopra. Ecco, cerchiamo di evitare di essere mosche che si schiantano sul vetro. Cito un rimedio, che non è mio. L'ex comandante del Comando supremo alleato della NATO in Europa, ammiraglio Stavridis, americano di origine greca, in un suo libro del 2017, commentando la situazione del Mediterraneo in relazione all'immigrazione e, in particolare, all'inazione dell'Unione europea di fronte ai problemi di Italia e Grecia, si chiedeva come mai l'Italia

che l'immigrazione di massa, così come l'abbiamo vista nel 2014, 2015, 2016 e 2017, era sicuramente un attacco e un problema di stabilità per il nostro Paese; ripeto,

a voler chiedere all'Europa qualcosa che non è disposta a dare, è evidente. Scusandomi per la digressione, concludo ribadendo il voto favorevole alle missioni internazionali,

ci ritiriamo dall'Afghanistan e prevalgono i talebani, è necessario probabilmente che i talebani diventino un problema per qualcun altro. Come dissi commentando il ritiro dall'Afghanistan, dopo l'audizione del ministro Guerini, sottolineo che oggi sono Cina e Russia ad avere un problema di stabilità ai propri confini, là dove i talebani dovessero acquisire maggiore forza in Afghanistan. Noi abbiamo un altro problema, che è il contenimento della potenza e prepotenza cinese, a partire dal Mar cinese meridionale e fino alle coste del Mediterraneo. *(Applausi)*.

mi rivolgo anche ai banchi del Governo estendendo il ringraziamento al sottosegretario Della Vedova, che hanno seguito i lavori delle Commissioni sia alla Camera che al Senato. Mi permetto di inviare un messaggio, che ho già avuto occasione di ribadire

in una riflessione seria sulle linee di indirizzo della politica estera del nostro Paese, di cui le missioni internazionali sono forse lo strumento più potente in termini di *hard power*, ma anche di *soft power* per la la componente di cooperazione allo sviluppo. Lo dico perché dobbiamo prenderci tutti l'impegno di discutere di missioni internazionali in anticipo. Da questo punto di vista, forse sarebbe necessaria anche una riflessione su quella legge, su come è costruita, sui tempi sulle modalità anche di trasformare veramente l'occasione del dibattito sulle missioni internazionali in una grande discussione sulle scelte di politica estera, sui nostri interessi strategici, sugli obiettivi che ci poniamo. Lo dico perché quando si parla di missioni internazionali bisogna

alla gestione di sfide complesse come quelle degli effetti più complicati della globalizzazione, come può essere la gestione dei flussi migratori; rifugiati che crescono nelle principali aree di tensione del Paese. Vale per la tutela degli interessi strategici del nostro Paese: va in questo senso il rafforzamento delle missioni sia nel Golfo di Guinea che nello Stretto di Hormuz, che si aggiunge alla missione Atalanta nello Stretto di Bab el-Mandeb. Vale per la grande sfida che non hanno gli altri Paesi fuori dal mondo occidentale e che abbiamo noi: quella di essere anche un faro per le democrazie liberali, ovvero quella della tutela dei diritti umani e dell'ambizione a far crescere gli *standard* di democrazia negli altri Paesi. Andiamo a insegnare la costruzione delle istituzioni nel momento in cui andiamo all'estero. Queste sono le grandi missioni che assegniamo alle donne e agli uomini delle Forze armate italiane, che voglio qui ringraziare a nome del Partito Democratico, insieme al ministro della difesa Guerini voglio segnare l'elemento di discontinuità forte che c'è stato negli ultimi mesi con la vittoria negli Stati Uniti da parte del presidente Biden, che ha riportato al centro del dibattito della comunità internazionale il tema del multilateralismo. Le missioni internazionali funzionano se i luoghi del multilaterale funzionano, e il messaggio che è partito dal G7, che si è recentemente concluso in Galles, è stato molto forte nel momento in cui Biden ha fatto la proposta, subito condivisa dai *partner* europei, del *build back better world.* Si tratta di un progetto molto forte in cui dice che non dobbiamo lasciare alla Cina e agli altri Paesi l'ambizione di essere un punto di riferimento a livello internazionale. Dobbiamo tornare a essere protagonisti nei diversi Continenti, in Asia, in Africa, ma non solo mettendoci i soldi per costruire le infrastrutture, non solo mandando i nostri uomini e le nostre donne nelle missioni internazionali, ma portando il peso della nostra storia e della nostra cultura, quindi la tutela dei diritti umani e *standard* di democrazia elevati. Questa è la differenza rispetto agli altri Paesi, e questo vale anche per il lavoro che dobbiamo fare con riferimento alle missioni internazionali. Dobbiamo riflettere anche sugli errori che sono stati fatti, perché l'amministrazione Trump ha rappresentato una regressione nella capacità di essere presenti in alcuni teatri internazionali. La vicenda dell'Afghanistan è sotto gli occhi di tutti. Sottoscrivo le parole del presidente Casini: abbiamo perso un'occasione. Abbiamo fatto un avanzamento dal punto di vista della tutela dei diritti umani del diritto delle donne. Avevamo proposto, per iniziativa della presidente Pinotti, una discussione e un approfondimento proprio su questi su questi temi. Voglio ringraziare il Ministero della difesa, il ministro Guerini in particolare, per l'attenzione rispetto alla comunità delle persone che hanno collaborato con noi in Afghanistan. Noi li riportiamo indietro e li tuteliamo, perché abbiamo la responsabilità di non lasciarli da soli in quel posto, esposti alla vendetta dei talebani. Ecco, da questo punto di vista si vede la differenza tra un grande Paese come l'Italia, che si fa carico della tutela dell'incolumità delle persone che hanno lavorato con noi, e un altro Paese. Questo vale anche in Iraq, dove stiamo spostando il nostro impegno dalla coalizione internazionale contro Daesh, a un impegno maggiore all'interno delle strutture NATO, proprio per far crescere la consapevolezza, la capacità e le *skill* delle forze di sicurezza irachene. Abbiamo un ruolo guida all'interno della missione NATO, che ci pone appunto al centro della capacità dell'Alleanza atlantica di essere protagonista in quell'area. È chiaro che questa esposizione dell'Italia deve avere un contrappeso e non possiamo che chiedere agli Stati Uniti, nell'ambito dell'Alleanza atlantica, un rafforzamento della strategia per il Sud del Mediterraneo, dove vi è l'esigenza l'esigenza di tutelare la maggioranza dei nostri interessi strategici: vale per il Mediterraneo orientale e vale per il Libano, che da un anno sta conoscendo una crisi senza precedenti.

delle istituzioni e della classe politica libanese di dare un governo stabile. L'Italia si trova da anni alla guida dell'operazione UNIFIL e riesce ad essere forse l'unico interlocutore anche per le forze politiche e sociali di quel territorio e dobbiamo essere orgogliosi della guida del comando italiano. Poi c'è il tema, più in generale, del Mediterraneo centrale. Lo voglio dire anche a chi ha espresso legittimamente preoccupazioni rispetto alla situazione in Libia: il Partito Democratico è impegnato in prima fila, perché conosce la situazione sul territorio, conosce la situazione drammatica dei campi di detenzione dove vengono calpestati i più elementari diritti umani, ed è impegnato a garantire l'aumento dei corridoi umanitari, la modifica del Memorandum d'intesa con i libici. Ma allo stesso tempo ha la consapevolezza e la certezza che lasciare al proprio destino la Libia sarebbe condannare quelle persone a un destino sicuro, in maniera analoga a quanto sta accadendo in Afghanistan. *(Applausi)*. Non ci possiamo permettere una Somalia alle porte di casa. Allora dobbiamo affrontare quelle contraddizioni, sporcarci le mani. È questo che fa la politica: affrontare i nodi, provare a risolvere le questioni che riguardano i campi di detenzione, aiutare il dialogo politico. Come possiamo aiutare il dialogo politico, per far sì che questo Governo di transizione debole arrivi alla fine e alle elezioni del 24 dicembre? Lo facciamo ritirandoci, o lo facciamo stando dentro quelle contraddizioni, affrontandole, certo attirandoci anche alcune critiche? Proviamo a farlo e lo facciamo con gradualità. Abbiamo convinto gli altri Paesi europei con noi a investire finalmente nell'operazione Irini, a dargli i poteri e le attribuzioni, e a far sì che dall'anno prossimo potranno fare loro direttamente la formazione e l'addestramento della Guardia costiera libica, in modo tale che non ci sia solo l'Italia, che essendo a pochi chilometri dalle coste può subire l'influenza di quel Governo. Ma non è da sola l'Italia, perché sarà insieme agli altri Paesi europei, sarà insieme all'Alto rappresentante nel poter tutelare i diritti umani e chiedere un innalzamento degli *standard*. La stessa cosa può essere fatta sul territorio libico. Noi abbiamo una grande ambizione: dare all'Europa - questa vuole essere la conclusione del mio intervento

Sono molto pragmatici. Loro sono al nostro fianco se anche noi ci sporchiamo le mani, se dimostriamo di farci carico di un pezzo della sicurezza globale. Non lo possiamo fare singolarmente. Lo abbiamo visto in Libia. in Libia si va ognuno per la propria parte - l'Italia, la Francia, la Germania - non otteniamo risultati. Noi, infatti, abbiamo scritto nella nostra Costituzione che non andiamo a fare la guerra e non mandiamo soldati, l'un contro l'altro armati, nelle guerre civili. Questa è una questione molto importante, perché noi siamo rispettosi di ciò che è scritto nella nostra Costituzione, ma non stiamo a guardare.

può contare quanto la Turchia, la Russia e gli altri attori che giocano un ruolo importante in Libia. Noi abbiamo investito in professionalità, in persone, in legami culturali in Libia: non perdiamo questa occasione. Chi scappa dai teatri difficili e complicati e non affronta le contraddizioni di quei territori ha solo da perdere e rischia di lasciare da sole quelle persone. Tra il velleitarismo e la *Realpolitik* cinica noi chiediamo di essere presenti in quel territorio con la tutela dei diritti umani, con la condivisione della responsabilità e con la serietà dell'impegno delle nostre donne e uomini delle Forze armate.

l'intervento delle anime belle, ma pone e ha posto anche nella discussione in Commissione una serie di questioni che sono, a mio avviso, assolutamente fondamentali, proprio in nome di quella Costituzione, che noi richiamiamo e che ho sentito richiamare anche negli interventi che mi hanno preceduto. preceduto. Tutti noi siamo assolutamente convinti che il nostro Paese debba aiutare la transizione in Libia che debba aiutare, col nuovo esecutivo di transizione, una stabilizzazione: non solo perché questo è l'interesse del nostro Paese, ma perché questo è l'unico modo per poter avere un'influenza vera all'interno dello scenario in Libia. Proprio per poter facilitare e sostenere una transizione verso una una situazione di assetto più democratico, a maggior ragione il nostro Paese, proprio in nome di quei valori della Costituzione, deve compiere delle scelte ben precise. Tornerò sulle questioni che riguardano tutto lo scenario del Mediterraneo, perché io condivido molto alcune preoccupazioni che sono state prima esposte. Io penso, però, che noi non possiamo più

anche delle convenzioni internazionali. Stiamo parlando, tra l'altro regolarmente, di respingimenti collettivi e sapete perfettamente che questi sono vietati anche dalle convenzioni internazionali. Gli organismi hanno decretato, in modo molto chiaro, tra l'altro, la Libia non è certamente un porto sicuro. Quindi, il ruolo che la Guardia costiera assume (e che noi, appunto, finanziamo) è evidentemente quello di continuare a riportare queste persone all'interno dei centri di detenzione. È un circolo vizioso, che noi finanziamo, perché noi finanziamo i centri di detenzione, per le spese sanitarie e per l'assistenza medica. Ma noi non abbiamo mai chiesto conto di come in realtà queste risorse, i nostri soldi, i soldi dei contribuenti italiani

in questi centri di detenzione ormai è acclarata. Non è che possiamo far finta di non vedere; non possiamo più far finta di non vedere. Il finanziamento arriva al paradosso che la motovedetta che abbiamo dato ai libici è quella che ha sparato; però tutti quanti a levare gli scudi contro i pescherecci italiani. Questa è la situazione. Nel conflitto per bande e per tribù che si è scatenato tra le milizie dopo la caduta di Gheddafi è

trafficanti di esseri umani. Questo è il punto. Qui non si tratta di essere noi le belle anime e gli altri quelli che si vogliono sporcare le mani, perché comunque devono aiutare le persone; qui si tratta di assumere delle decisioni e quindi di sospendere quella missione, altrimenti rischiamo continuamente, ogni giorno, di essere complici di una violazione sistematica

Ogni anno viene reiterata la stessa promessa; quest'anno la promessa è che questa volta coinvolgeremo l'Europa. Ma non cambia; non è che, se non sarà solo l'Italia, ma sarà l'Europa a continuare a far finta di non vedere, le cose cambiano. Credo che questo non ce lo possiamo più permettere. Per questo motivo noi chiediamo - l'abbiamo già chiesto, l'ha chiesto la collega

perché abbiamo visto documenti, rapporti e immagini video di quello che succede. E io credo che un Paese come il nostro non possa fare questo. Diceva il collega Verducci che l'Italia deve tornare lì a fare l'Italia; a fare l'Italia; e fare l'Italia significa essere noi i portatori dei nostri valori, della difesa dei diritti umani e non dire genericamente che ci preoccuperemo e che vedremo cosa accade nei centri di detenzione. Questa storia si è ripetuta continuamente a ogni rinnovo

capire la vicenda dell'Afghanistan e tutte le altre questioni. Vi è la preoccupazione del Mediterraneo: dovunque guardiamo nel Mediterraneo (vogliamo fare l'elenco dei Paesi?)

dei confini e dell'immigrazione, sbagliando tutto, perché poi non si controlla nulla - questi sono gli errori - senza la capacità di esprimere una *leadership* su quello che sta accadendo in tutti questi Paesi. di situazioni molto preoccupanti, che rischiano di consegnarci uno scenario non più certamente gestibile, oltre il conflitto, oltre quello che sta accadendo e chi

e riflettere, una volta per tutte, su cosa significa pensare di esportare la democrazia. Questo è il risultato! Quella è stata, alla fine, un'operazione fallimentare e i risultati saranno tremendi per la popolazione.

di altri colleghi, che non hanno avuto modo di parlare. Francamente però arrivo soltanto a capirli, ma non condivido le loro perplessità e cercherò di argomentare questa mia non condivisione, favorevole, che già annuncio, alle due risoluzioni da parte del MoVimento 5 Stelle, partendo da una considerazione che credo sia condivisa da tutti in quest'Aula, ossia che in politica estera il concetto di vuoto non esiste. Il concetto di vuoto, in questo senso, è inteso come l'assenza di attori di rilievo negli scenari internazionali,

tale esempio è già stato riportato a proposito della mancanza di un attore importante, come gli Stati Uniti d'America, durante la presidenza Trump (e si spera non anche durante la presidenza Biden) nello scenario mediorientale e nello scenario del Mediterraneo allargato.

La mancanza di una presenza forte ha portato alla situazione che abbiamo visto negli ultimi otto o dieci anni, che è stata descritta da numerosi colleghi, compresa l'ultima collega intervenuta, la senatrice De Petris. Le missioni internazionali sono, per l'Italia, il principale strumento dell'esplicitazione della politica internazionale, intesa proprio con le caratteristiche che il nostro Paese ha sempre mantenuto all'interno degli scenari internazionali. Cito prima di tutto, tra tali caratteristiche, proprio quella di fare ogni cosa affinché non vengano lasciati dei vuoti negli scenari di prossimità e, soprattutto, negli scenari rilevanti per la sicurezza internazionale. La seconda caratteristica della politica internazionale italiana è quella di riuscire a operare, soprattutto di crisi, con le caratteristiche proprie e particolari della nostra tradizione di politica estera. Sono diverse le missioni internazionali di cui ci siamo occupati, ma prenderò a riferimento soltanto alcuni esempi. Il primo esempio Il primo esempio è proprio quello citato da molti colleghi, ovvero il rinnovo della missione di assistenza alla guardia costiera libica da parte del nostro Paese. Su questo si sono espressi in tanti ed io vorrei riprendere in in parte le parole della senatrice Rauti, che ha detto a un certo punto che in Libia non ci vogliono e magari preferiscono altri e sarebbe preoccupante se questa preferenza fosse soprattutto per i turchi.

non mi sembra che non ci vogliano. Se l'ansia di Fratelli d'Italia è di fare opposizione a tutti i costi, la facciano pure, ma non mi pare che sia questo il caso. Il ruolo della politica estera italiana è quello che io ricordavo e che mi piace ribadire ancora una volta, e cioè essere attori particolari come lo siamo in Libano.

con gli islamici; arriva a parlare con Hezbollah, considerata una formazione terroristica. Ma se non ci fosse il contingente italiano, immaginiamo per un momento che cosa succederebbe in quel teatro. Accadrebbe la stessa cosa che accadrebbe se l'Italia abbandonasse la missione a sostegno della guardia costiera libica: qualcun altro andrebbe a colmare quel vuoto. Non nego che in Libia ci siano fazioni che governano pezzi dell'apparato di sicurezza o delle forze militari, ma quello che è impossibile da realizzare oggi nel contesto che stiamo vivendo è abbandonare la Libia al proprio destino. Ed è quello appunto che non stanno facendo i nostri rappresentanti di Governo, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, prima fra tutti la politica dei vaccini. Dare la possibilità possibilità non solo alla Libia, ma anche alla Tunisia di avere dosi vaccinali che arrivano in dono dall'Italia è sicuramente un punto a sostegno della nostra presenza in Libia. Del resto, lo abbiamo visto: se non ci fosse questo tipo di politica, il vuoto sarebbe colmato da altri, così come ha fatto appunto la Turchia durante i mesi tristi e bui del conflitto tra le due fazioni di Tobruk e di Tripoli.

per la stessa logica con la quale negli anni 1987-1988, in pieno conflitto tra Iran e Iraq, il ministro degli esteri di allora, Giulio Andreotti, incontrava il ministro degli esteri della Repubblica islamica iraniana Ali Velayati più e più volte a Fiumicino. Lo ricordo, lo scrivevano i giornali italiani, ma me l'ha ricordato lo stesso Velayati, che ho incontrato nell'aprile del 2019, durante una missione ufficiale autorizzata dalla presidente Casellati in Iran, a testimonianza di quel modo particolare di fare politica estera italiana. E questo modo particolare è quello di essere presenti senza pregiudizi in tutti gli scenari e lo faceva Giulio Andreotti da Ministro degli esteri incontrando Velayati a Fiumicino. Velayati perdeva cinque ore prima di recarsi a New York all'Assemblea delle Nazioni Unite per scambiare con Andreotti impressioni questo me l'ha raccontato Velayati - che l'Italia non poteva avere se non da un confronto diretto e ricevere dal Ministro degli esteri italiano impressioni che quella parte del mondo non avrebbe potuto ricevere Poi naturalmente Andreotti riferiva agli alleati occidentali, come è giusto e doveroso che fosse. Tuttavia, contrariamente a quanto alcuni colleghi in quest'Aula hanno ribadito più volte, non c'era assolutamente una una chiusura nei confronti del dialogo con un Paese che già allora era considerato pericoloso per la stabilità internazionale, tant'è che in quei mesi gli Stati Uniti bombardarono le piattaforme petrolifere proprio al largo dello Stretto di Hormuz e nello stesso tempo il nostro Paese dialogava con i rappresentanti politici della Repubblica islamica dell'Iran. Questo è il modo italiano di fare politica estera e lo dobbiamo ribadire ancora una volta, perché io ritengo che oggi il nostro Paese debba essere saldamente ancorato nelle alleanze economiche e militari, saldamente parte del processo di riunificazione (in senso vero) dell'Unione europea, ma non deve perdere quelle caratteristiche che ne hanno fatto una media potenza che ha saputo dialogare nel tempo anche con chi non era vicino ai propri interessi nazionali. in questo momento, ribadendo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alle due proposte di risoluzione, vada sottolineata soprattutto la lunga e sana tradizione della politica estera italiana

hanno chiesto la votazione per parti separate, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, della scheda n. 48 relativa al Documento

che prevede la votazione per parti separate delle schede nn. 48, 18, 34 e 47, che verrebbe preclusa nel caso di approvazione della richiesta della senatrice Bonino. Qualcuno è contrario?

nuova finestra"). Senatore Ciriani e senatore Bruzzone, riferisco rispetto alla richiesta di riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

«Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa». Pertanto, da questo momento fino ad allora

tutte le forze parlamentari intervenute in dissenso da una nomina completamente sbagliata di una persona vicino alla famiglia Benetton e Castellucci, che ha portato alla tragedia del ponte Morandi, ha ritirato la propria candidatura e si è dimesso di fatto. *(Applausi)*. Si riapre la discussione e vorrei ringraziare tutti perché oggi il Parlamento è stato completamente vicino a Genova e a tutte le famiglie

colleghi, i cambiamenti climatici repentini, improvvisi e anomali stanno mettendo in ginocchio le coltivazioni agricole in molte parti del nostro Paese. Il nostro territorio è segnato da continue, pesanti e violente grandinate, piogge torrenziali e vento forte che finora hanno mandato in fumo migliaia di ettari di colture e decimato - in alcuni casi dimezzato - la produzione agricola. La stima dei danni nella sola provincia di Cuneo ammonta a oltre 19 milioni di euro, tra produzioni e strutture, per un totale di 6.000 ettari di colture duramente colpite. A farne le spese sono soprattutto il mais, i cereali, la frutta, le verdure e la vite. Il resoconto dei danni della grandine ha coinvolto molte zone dal Saluzzese, al Monregalese, al Fossanese - e in interi territori, come nei Comuni di Vottignasco, Levaldigi e Villafalletto, sono stati necessari trattori con le pale per pulire le strade dalla grandine. È stata colpita anche una parte importante della città capoluogo. Quello che più stupisce di questi fenomeni atmosferici è come colpiscano a macchia di leopardo: può succedere così che un campo riporti danni del 10 per cento e in quello successivo, a pochi chilometri di distanza, distanza, superino addirittura il 50 per cento. È un'estate, quella italiana, segnata fino ad ora a livello nazionale da ben 789 eventi estremi, tra bombe d'acqua, trombe d'aria, grandinate, temporali violenti lungo tutta la penisola. Sono praticamente triplicate le grandinate, con undici tempeste di ghiaccio al giorno dall'inizio dell'estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa situazione ormai non può più essere trattata come una semplice emergenza, dal momento che si innesta su eventi ormai continui di vere e proprie bombe d'acqua rapide e violente. Per affrontare i danni causati dagli eventi estremi servono strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, di semplice accesso per le nostre imprese agricole, efficaci e con meno burocrazia, che prevedano risarcimenti immediati secondo tempistiche certe per aiutare i nostri agricoltori a risollevarsi. Noi facciamo appello al Governo perché intervenga immediatamente attivando il Fondo di solidarietà nazionale e mettendo le risorse a disposizione della Regione. Una proposta da parte del nostro Gruppo potrebbe essere il rifinanziamento mirato dell'istituto della cambiale agraria di Ismea solo per chi ha subito danni fino a 50.000, a tasso zero per sette anni, con due anni di preammortamento. Questo potrebbe essere uno strumento immediato, già conosciuto e di facile accessibilità. Diamo risposte immediate, poiché i nostri agricoltori non possono più aspettare. *(Applausi)*.

riguarda le condizioni a dir poco assai critiche dell'assistenza sanitaria nella vasta area del golfo di Policastro, a sud di Salerno. L'ospedale di Sapri, incardinato nella ASL Salerno 1, serve questo vasto territorio prestando assistenza sanitaria ai numerosi paesi che si affacciano sul golfo stesso. In questo periodo, sulla costiera cilentana è presente un milione circa di turisti. Queste presenze così ragguardevoli di turisti evidentemente portano a un aumento esponenziale della domanda di servizi e prestazioni sanitarie. Senonché le autorità regionali che dovrebbero provvedere a ciò - com'è noto, l'articolo 117 della Costituzione affida alla Regione la competenza per la materia dell'organizzazione sanitaria - sono evidentemente prese da tutt'altri pensieri. Si legge sulla stampa di oggi che il governatore De Luca è tutto preso

Si pensi che l'organico di diritto dei cardiologi, di circa dieci unità, è ridotto di fatto a quattro sanitari soltanto, i quali stanno conducendo attualmente turni orari ore al giorno. L'ospedale sta collassando. Lo stesso dicasi per chirurgia, ortopedia e pronto soccorso, che sono i settori più incandescenti nel periodo estivo a causa di incidenti, traumi e quant'altro. Questa situazione molto grave non è di oggi, ma è diventata strutturale e cronica, e non è mai stato fatto nulla per risolvere i paurosi vuoti di organico.

che definisce il diritto alla salute un diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività e ne affida la tutela - attenzione - alla Repubblica cui, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, si intende lo Stato ordinamento, tutti i poteri dello Stato. Quindi, non è inappropriato che ne parliamo in questa sede. signor Presidente, con una manifestazione di solidarietà per il Comune di Sapri, per i medici e gli infermieri che si stanno sacrificando fino allo stremo per il Comitato di lotta permanente, che costituisce espressione diretta di quelle comunità, affinché la loro lotta possa raggiungere l'obiettivo prefisso, che è quello di risvegliare dal letargo le autorità sanitarie regionali.

la vicenda Monte dei Paschi di Siena. Sarò breve, con una cronistoria veramente lampo su una vicenda che sta suscitando grande preoccupazione sicuramente nella città di Siena e in Toscana, ma oggettivamente anche in Italia e sui mercati internazionali. Nel 2018 il Partito Democratico candida nel collegio di Siena l'ex ministro Padoan, che viene eletto deputato della Repubblica. Qualche mese dopo - perché di questo si tratta - l'ex ministro e quindi deputato e, di lì a poco, ex deputato del Partito Democratico si dimette e diventa presidente di Unicredit.

Unicredit si lancia verso la banca, che nel frattempo aveva ottenuto 5,4 miliardi dallo Stato per non fallire; se ne chiede uno sconto fiscale per l'acquisizione. Insomma,

Forza Italia è stata la prima a denunciare la questione, a livello sia locale che nazionale, e vogliamo ribadirlo anche nell'Aula del Senato. Noi non ci fermiamo: non consentiremo questo saccheggio, non consentiremo ancora una volta alla sinistra italiana, al Partito Democratico, di portarsi a casa una banca, come ebbe a dire Fassino a Consorte: «Ma abbiamo una banca?». Detta roba, questa volta, non la consentiremo nella maniera più assoluta, nell'interesse dell'Italia, nell'interesse di Siena, della Toscana e di un mondo che ci guarda francamente sopraffatto da un fatto che soltanto, probabilmente, nel nostro Paese può accadere.

vorrei stigmatizzare l'ennesimo episodio di violenza e di aggressione - in questo caso per fortuna solo verbale - subìto dal personale sanitario medico e infermieristico, avvenuta a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli; oggetto delle minacce verbali è stato il personale del 118, presente su un'autoambulanza impegnata nel primo soccorso. Ebbene, due giovani in *scooter* hanno affiancato il mezzo di soccorso, sferrando pugni e calci al veicolo, apostrofando gli operatori a bordo dello stesso con offese verbali, epiteti e minacce, con un linguaggio aggressivo e volgare. «Se passi di qua devi chiudere queste luci»: questa è la fase imperiosa e minacciosa quasi ad affermare il loro personale potere di concedere o meno il permesso di attraversare quel territorio, quasi fosse il loro territorio, probabilmente perché i lampeggianti dell'autoambulanza si potevano confondere con quelli della polizia. Questo è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo, ma certamente non resterà tale, di aggressione subìta dai medici e dal personale sanitario del 118, ma in generale di tutta l'area dell'emergenza, compresi i pronto soccorso ospedalieri e le guardie mediche, che sono ripetutamente oggetto di aggressioni e sottoposti a enormi stress psicofisici, ancor di più in questo periodo di emergenza pandemica. Questa situazione è anche legata a una cattiva organizzazione, particolarmente sentita in alcuni territori dell'area dell'emergenza territoriale, che necessita di una completa e attenta riorganizzazione. La collega, senatrice Castellone, a tal proposito ha presentato un disegno di legge che, con il contributo di tutta la Commissione sanità, pur nelle differenti sensibilità e posizioni politiche presenti, dovrà necessariamente portare a una riforma del 118 e più in generale della rete dell'emergenza-urgenza, non più procrastinabile. Non basta chiamare semplicemente a parole "eroi" i medici e gli operatori sanitari che operano con impegno ed abnegazione tutti i giorni, rispondendo alla domanda di emergenza salute,

Signor Presidente, colleghi, nel film «Totòtruffa '62», a tutti noto, il cavaliere Antonio Trevi, asserito discendente dei proprietari dell'omonima fontana, intavola con l'oriundo-americano Decio Cavallo una spassosissima trattativa per l'acquisto della fontana del Bernini. Il prezzo pattuito è 10 milioni, ma la caparra che Decio Cavallo verserà, grazie anche all'intervento del cavaliere Scamorza, Nino Taranto, presunto concorrente nella compravendita, ammonta a 500.000 lire, cifra all'epoca considerevole. È così che il povero Decio Cavallo non solo ci rimette mezzo milione, ma sarà portato via con la forza dai sanitari che lo credono matto, perché si proclama proprietario della Fontana di Trevi. L'intero film, articolato in più episodi, è un inno all'italianissima arte di arrangiarsi, messa in atto dai furbi a spese degli ingenui, esasperata volutamente fino al paradosso. Questa truffa in particolare, però, è rimasta celebre anche perché coinvolge uno dei monumenti simbolo di Roma; anzi, se escludiamo la Basilica di San Pietro, forse il monumento per eccellenza dopo il Colosseo. Sessant'anni fa Castellano e Pipolo, gli autori del soggetto, non osarono immaginare che Totò e Nino Taranto potessero addirittura vendere il Colosseo; ma, se avessero potuto assistere, il 28 agosto scorso, alla sceneggiata allestita per il G20 Cultura nell'arena dell'Anfiteatro Flavio, si sarebbero inchinati davanti a uno sceneggiatore e regista, l'onorevole ministro Franceschini, che, grazie a un talento naturale per il comico, anzi per il farsesco, ha osato l'impensabile: esibire e vendere il Colosseo ai venti grandi sprovveduti della terra. Dopo non li hanno portati via per il TSO, per cui probabilmente ignorano tutt'ora di essere i Decio Cavallo di turno, oggetto di una truffa clamorosa, ordita appunto dal Ministro della cultura, che si è fatto passare per il proprietario del monumento, anche grazie alla spalla comica offertagli dal Presidente del Consiglio. In Costituzione il patrimonio culturale appartiene al popolo a titolo di sovranità, non certo al vertice politico come strumento di promozione personale, né alla pubblica amministrazione, che tuttavia l'ha in consegna per conto dei cittadini per realizzare il mandato costituzionale prioritario di tutelarlo e conservarlo; quello che dovrebbero fare gli archeologi, gli inutili esperti che Draghi ha sconfessato nell'ignobile siparietto finale con Franceschini. Si tutela e si conserva un monumento, non per esibirlo come sfondo nelle foto ufficiali né per farne una macchina da soldi da regalare agli speculatori, ma perché esso va conosciuto e compreso da tutti; perché appartiene alla storia e dunque ha il compito di ammonire (*monumentum* vale ammonimento); perché deve favorire lo sviluppo morale e spirituale degli individui affinché siano più consapevoli e attivi anche come cittadini. Non è di poco conto quello che è successo il 28 luglio e le dimissioni dei due disonorevoli sarebbero state richieste da tutte le forze politiche in un Paese sano. Aggiungo, signor Presidente, che da stamane il Parco del Colosseo pubblicizza l'ingresso a pagamento per i cittadini proprietari dell'area monumentale che vogliano all'alba praticare attività fisica entro i confini dell'istituto. Siamo alla prostituzione di Stato. I romani pagheranno per accedere a uno spazio che è già loro, che si mantiene anche con le loro tasse e che già pagano, al pari degli altri visitatori, per entrare nell'anfiteatro: 12 euro di base più 2 di prenotazione obbligatoria più 4 di mostra obbligatoria. Presto pagheranno, pagheremo, per poterlo fissare senza distogliere lo sguardo. la ringrazio della cortesia di avere ammesso il mio intervento. In realtà, io intervengo per un fatto importante che riguarda un nostro connazionale, un diplomatico, un friulano un uomo della mia terra, che è stato per oltre vent'anni all'ONU. Ambasciatore, Vice Segretario Generale dell'ONU, ha contribuito alla liberazione di diversi ostaggi ed un soldato disarmato della democrazia nel mondo. Oggi Giandomenico Picco, friulano, figlio di un farmacista e di una casalinga, si trova negli Stati Uniti, affetto da una grave forma di Alzheimer. informazioni di amici, che non abbia le sufficienti cure. Noi riteniamo che il nostro Paese debba intervenire. In questo senso la comunità friulana si è mossa. Si è mosso il Presidente del Consiglio regionale si sono mosse diverse personalità. Noi vogliamo riportarlo in Friuli, dove gli assicureremo le cure necessarie. Noi riteniamo che egli meriti quel riconoscimento che si chiama legge Bacchelli, che viene concesso ai cittadini italiani illustri.

confido nella sensibilità del Governo e nella sensibilità del Parlamento affinché si trovino le forme, i mezzi e i modi necessari per assicurare a Giandomenico un ritorno in patria decoroso e dignitoso.